Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3*-ter* del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 981 «Bilancio di previsione dello Stato

In conformità all'articolo 161, comma 3*-ter* del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento, nonché alla luce del parere della 5aCommissione permanente - cui l'emendamento viene immediatamente trasmesso - ai sensi del combinato disposto degli articoli

trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - i commi da 160-*bis* a 160-*novies* dell'articolo 1 siano soppressi; al comma 421 dell'articolo 1, le cifre ivi indicate siano sostituite con quelle indicate, in riferimento al medesimo comma, dalla Relazione tecnica; - al comma 653 dell'articolo, le cifre ivi indicate siano sostituite con quelle indicate, in riferimento al medesimo comma, dalla Relazione tecnica; con le seguenti osservazioni: - i commi 163-*octies* e 163-*novies* dell'articolo 1 dovrebbero essere espunti, in quanto non compatibili con il comma comma 187-*quaterdecies* del medesimo articolo; - al comma 167-*bis* dell'articolo 1, per un errore materiale, non sono state allegate le tabelle I e II che il Governo deposita in seduta e di cui sono a disposizione le copie; il comma 429-*bis* dell'articolo 1, per un errore materiale, viene riprodotto tre volte, per cui occorre rinumerare come *ter* la seconda disposizione e sopprimere la terza, che è identica alla precedente; l'emendamento reca, alle pagine 189 e seguenti, una serie di modifiche alla II Sezione del disegno di legge, che andrebbero espunte, per un'esigenza di coordinamento con gli identici emendamenti approvati dal Senato nella seduta di ieri. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo accolgo le condizioni e le osservazioni formulate dalla 5a Commissione permanente che entrano a far parte integrante del testo. Onorevoli colleghi, alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e dell'intervento del Governo, la Presidenza ritiene ammissibile l'emendamento 1.9000, come riformulato.

Presidente, io credo che, forse, si doveva quantomeno contestualizzare cosa è successo poc'anzi in Commissione bilancio.

Signor Presidente, lei sta avallando dei *vulnus* nei confronti del Parlamento che sono sempre più gravi. Tutte le minoranze

con violenza, ha lavorato affinché il Senato non potesse leggere questa manovra, che è ricca di cose molto gravi per il Paese! Allora, signor Presidente, faccia la Capigruppo, ma non credo che nel rispetto dell'articolo 72 della Costituzione si possa procedere alla votazione come se nulla fosse. Ogni minuto c'è un'offesa in più, c'è una ferita in più nei confronti della democrazia. Lei e il Senato vi dovete opporre!

Diteci che cosa state tenendo nascosto agli italiani. Fateci vedere Basta con questi giochi di prestigio sulla pelle degli italiani. Signor Presidente, ieri abbiamo avvertito il Governo

tutti quegli elettori che hanno creduto nella maggioranza e che questa manovra potesse avere un significato. Questo è un fallimento politico, lo sappiamo; non vogliamo dire Caporetto? Diciamo Waterloo. Presidente, abbiamo cercato di difendere la maggioranza da se stessa. Mi fa piacere che voi siate così ilari. È bello che il pensiero di ridurre gli italiani in mutande vi diverta tanto. Bravi! Complimenti! Vogliamo vedere una manovra che purtroppo si annuncia di tagli, di tasse, di tanta IVA e di clausole di salvaguardia che scatteranno e purtroppo ogni giorno non è quello giusto.

Non mettete questo Parlamento ulteriormente in difficoltà nei confronti del Paese. Colleghi, amici, la figuraccia la stiamo facendo tutti, e non solo voi che gestite questa manovra in maniera dilettantesca.

dai Gruppi FI-BP e PD)*. Commissioni che si convocano, che si sconvocano, *streaming* negati: ma di che cosa avete paura? Questo Governo si compone anche di una forza politica che faceva della trasparenza e dell'apertura del Parlamento come una scatoletta di tonno la sua cifra distintiva. Amici, vi è scappato il tonno! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Anziché una scatoletta di tonno aperta, volete farci approvare questa manovra a scatola chiusa. Noi non ci stiamo. Signor Presidente, chiediamo ancora una volta - ce ne dispiacciamo e ce ne vergogniamo un po', anche se non è colpa nostra, perché i ritardi non sono colpa nostra, li stiamo subendo esattamente come il popolo italiano e li pagheremo sulla nostra

dei Capigruppo perché denunciamo qui quello che è accaduto in Commissione bilancio: c'è una violazione chiara e precisa

il destino del Paese: carta vince, carta perde. Mettono delle norme, poi le tolgono; non vogliono dare spiegazioni; nella relazione tecnica c'è scritto altro. Le ricordo, Presidente - ma lei lo conosce meglio di me - l'articolo 161, comma 3*-quater*, del Regolamento: «Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo». Non può

interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 981 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che recepisce le condizioni e le osservazioni formulate dalla 5a Commissione permanente

La Conferenza dei Capigruppo ha nuovamente rimodulato i tempi della discussione sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo della prima sezione della legge di bilancio, spostando le dichiarazioni di voto finali alle ore 23,30 al fine di consentire lo svolgimento della discussione nei tempi già definiti ieri, vale a dire circa tre ore e trenta minuti. Pertanto la diretta televisiva avrà luogo nel nuovo orario delle 23,30.

comincio dalla fine questa volta. Ci sembra, dopo quello che è successo oggi in Commissione, una rottura totale dello spirito costituzionale e democratico: numeri sbagliati, conti che non tornano, stralci, presidenti barricati dentro la Commissione, oltretutto sempre di quel movimento politico che faceva della trasparenza, dello *streaming*, come dicevamo prima,

proprio di quel movimento politico che dianzi menzionavo, in una sua famosa manifestazione a Bologna nel 2007, il famoso Vaffa day. Non ne possiamo più. Ma il problema, signor Presidente, è che loro stanno mandando a quel Paese gli italiani! Questa è una presa in giro nei confronti degli italiani! stanno imbavagliando noi, che abbiamo chiesto di poter votare domani mattina, chiedendo le dichiarazioni di voto e il voto finale in diretta televisiva domani mattina. Ancora una volta, di che cosa avete paura? Avete paura che si veda il contenuto di questa manovra, che sarà di lacrime di sangue per gli italiani? Avete paura che gli italiani la domenica mattina se ne accorgano? Non volete turbare la loro sensibilità? *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Noi voteremo alle 23,30. Anzi, no, molto più tardi. Alle 23,30 comincerà la diretta televisiva. Quindi, noi voteremo alle 2 di notte. E chi si aggira di notte, a parte la Befana? Chi si aggira alle 2 di notte a parte a parte la Befana, viste le festività natalizie? Quelli che entrano di nascosto nelle case degli italiani. *(Applausi di farvi giudicare dagli italiani. Voi, quelli dell'onestà! Voi, quelli della trasparenza! Voi, quelli dell'*hashtag*: streaminglaveritàpertutti! Non avete il coraggio di far sentire la voce delle minoranze prima delle 2 di notte! e PD)*. State rendendo un servizio infame alla democrazia. Non abbiamo più parole per dirvi quanto orribile sia questo comportamento parlamentare. Ancora una volta, mi suggeriscono: sconcio. Avete paura di dire che pagherete il reddito di cittadinanza con i soldi dei pensionati che guadagnano 1.300 euro al mese, dopo una vita di lavoro? Avete paura: ditelo! Non ditelo alle 2 di notte! Abbiate il coraggio di dirlo alla luce del sole, non come i ladri di notte o come la Befana! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Gli italiani si troveranno un pacco di Natale molto doloroso e molto vuoto sotto l'albero. Avete paura di dire che avete tagliato tutti gli incentivi possibili e immaginabili a quelle categorie produttive cui avevate promesso tutto: agli artigiani, ai commercianti, alle partite IVA e agli imprenditori. Avete tolto loro la vita! Avete paura di dirlo? Abbiate il coraggio delle vostre azioni. Non fateci votare alle 2 di notte. Ricordatevelo: gli italiani lo capiranno. Lo sapranno comunque! Noi che abbiamo spirito democratico siamo rimasti qui fino alla fine, ma non ve la perdoneremo. Non ve la perdoneremo! E faremo fino in fondo la nostra

una speranza è quasi un periodo ipotetico dell'irrealtà - in un ravvedimento operoso ed attivo. Speriamo che ci mettiate in condizione di farci sentire dal Paese quando diremo le nostre verità, che evidentemente sono più forti delle vostre se non ce le volete far raccontare. Speriamo che si voti domani mattina. Speriamo che gli organi di informazione trasmettano queste cose, anziché continuare a dire che non esiste opposizione. L'opposizione c'è! Dateci voce! Fateci sentire! Dateci voce! Noi ci siamo e lotteremo fino alla fine, perché voi dovete rendere conto di questo scempio agli italiani. Da adesso in poi, noi ci saremo sempre!

a dimostrazione della considerazione che ha già mostrato in questi mesi per il Parlamento e per il Senato della Repubblica. Capisco che nel periodo di Natale si fanno tante cene, c'è da comprare i regali e il ministro Fraccaro, come del resto il presidente

Il ministro Fraccaro, nella sua nuova veste non di Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma di burattinaio, si è seduto nell'anticamera del Presidente della Commissione bilancio, è andato personalmente a gestire i lavori

strumentalmente ha deciso di prendersi un'ora e trenta, delle due ore che nella Capigruppo avevamo deciso per approfondire il maxiemendamento,

Però, il presidente Pesco, che prima ha provocato e ha annunciato che avrebbe espulso chiunque l'avesse interrotto, in realtà aveva il suo piano: doveva far votare senza discutere. Complimenti, Presidente ha lavorato bene dietro la regia del ministro Fraccaro. Complimenti! Vede, signor Presidente, lo abbiamo studiato tutti a scuola: ci sono delle regole nella democrazia. Non possiamo e non dobbiamo accettare che l'Esecutivo, con il proprio Ministro per i rapporti con il Parlamento, venga a dettare la linea in Commissione. Non possiamo accettare che il Governo svolga anche la funzione del Senato, del legislativo. Ci dobbiamo ricordare della divisione dei poteri, caro signor Presidente. È per questo che il Partito Democratico, viste le gravissime violazioni dell'articolo 72, non del Regolamento, della Costituzione italiana, quella Carta alla quale tutti noi ci dovremmo ispirare, esprime la volontà di sollevare, come Gruppo parlamentare, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, il ricorso diretto alla Corte costituzionale, affinché il giudice delle leggi si pronunci sulle enormità

dei diritti del Parlamento e viene a fare prepotenze e ferite senza precedenti. È una cosa inaudita e siamo costretti ad andare alla Corte costituzionale per la prima volta nella storia storia della Repubblica, perché dovete conoscere la gravità di quello che state combinando contro il Paese e contro gli italiani!

Signor Presidente, devo dire che nella mia non breve carriera politica - ho frequentato aule meno prestigiose di questa - difficilmente mi è capitato di dire: «Non ho parole». In questa occasione devo dire che io personalmente e i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia siamo rimasti senza parole, perché lo spettacolo messo in scena da parte della maggioranza francamente è difficile da commentare rimanendo fedeli al dettato del rispetto istituzionale che noi dobbiamo a voi e voi dovete a a noi, Presidente e colleghi della maggioranza. Non voglio fare un intervento di politica - ne parleremo più avanti nel corso della serata e della notte - ma voglio fare un semplice discorso di metodo e di rispetto. Francamente, abbiamo acconsentito tante volte ai cambiamenti di programma da parte della maggioranza; abbiamo sempre atteso pazientemente che la maggioranza decidesse quando e come discutere, anche del maxiemendamento. Anche questa volta abbiamo ricevuto "pesci in faccia" rispetto alla nostra disponibilità e responsabilità. Se volessimo avere rispetto innanzi tutto di noi stessi, e del ruolo che svolgiamo per mandato popolare, dovremmo chiedere perlomeno due-tre giorni di esame in Commissione per capire almeno superficialmente cosa c'è scritto in quel pacco di maxiemendamento che soltanto oggi pomeriggio il Governo ha consegnato in Commissione. Tuttavia, ci rendiamo conto, noi forse prima della stessa questo significherebbe l'esercizio provvisorio, e noi abbiamo a cuore prima di tutto gli interessi del nostro Paese, prima ancora e forse addirittura di più di quanto non ne abbia la maggioranza, che ha dimostrato devo dire la verità - grave irresponsabilità e dilettantismo nella gestione di questa partita così importante. Faremo quello che la maggioranza chiede: ci chiede di stare qua tutta la notte? Staremo tutta la notte a discutere e a portare il nostro contributo, spero costruttivo, nonostante il muro che la maggioranza ha creato intorno al proprio maxiemendamento. Mi consenta soltanto - e ho concluso, Presidente - una piccola nota nei confronti del ministro Fraccaro, che adesso non è in Aula. Quando si è seduti in maniera così evidente dalla parte del torto, un Ministro della Repubblica, prima di alzarsi e chiedere la fiducia, con un tono - mi consenta - vagamente provocatorio, dovrebbe avere un minimo di intelligenza politica - lo dico senza alterigia,

e sicuramente il clima della discussione che ci aspetta sarebbe stato migliore. Invece, nonostante gli errori, si continua con un atteggiamento che o è provocatorio o ha bisogno di altra aggettivazione che devo risparmiarmi perché siamo nel Senato. Signor Presidente, invito quindi lei, i colleghi della maggioranza e il Governo a rendersi conto delle condizioni in cui siamo costretti ad operare. Noi manteniamo la linea della responsabilità, ma, mi creda, non è un'impresa facile.

rivela. Lei sa, Presidente, che tutti noi siamo qui tra l'esasperato e l'esausto;

indietro nel tempo. Ha fatto tutto la maggioranza, incapace di riuscire a farci lavorare in Commissione, a determinarsi, a dare un minimo di compostezza. Lo sappiamo tutti - ahimè - che cosa sta accedendo; dovremmo riflettere a lungo rispetto a cosa è diventata la prassi della fiducia, ma questa sarà una riflessione che tutti quanti dovremo fare pacatamente. però arrivati al punto in cui, nonostante tutto quello che è accaduto in queste settimane, che gli impegni presi in Commissione sono stati puntualmente traditi. L'ultimo impegno ieri era quello di avere almeno la possibilità di avere due ore. Presidente, due ore! Lei sa che anche nella proposta calendario che abbiamo fatto ieri avevamo chiesto, tra l'altro, di avere un po' più di tempo almeno in Commissione.

hanno fatto, ancora davanti alle richieste di avere le ulteriori modifiche presentate? Come si fa non pensare che come al solito era tutto prestabilito? Ovviamente la discussione, il Parlamento, le Commissioni sono di impiccio e di impaccio. Tutto per coprire ancora una volta l'incapacità a scrivere un maxiemendamento, a determinarsi. Peraltro, Presidente, in questo maxiemendamento, per quello che abbiamo potuto vedere, vedere, ci sono cose molto diverse anche rispetto a quelle che in qualche modo si erano adombrate. Noi ci troviamo con ulteriori tagli pesanti. Vogliamo parlare dell'ulteriore pesantissimo taglio agli investimenti? Che cosa significa questo? Questo è quello che esce da questo maxiemendamento. Menomale che la chiamavano una manovra espansiva: questa è una manovra ancora una volta recessiva e rigorista, che fa cassa nel solito

ancora una volta diventa un modo per prenderci in giro, anzi per impedire strumentalmente la possibilità di qualsiasi discussione. Si arriva con il parere; questa è una cosa,

non ha avuto la possibilità neanche di finire di leggere. Questo è veramente inaudito. Come si fa? Siamo andati tutti al Quirinale e abbiamo sentito le parole del Presidente della Repubblica, che non ha richiamato solo me o solo lei, ma tutti. Ha richiamato a ridare forza e a rimettere al centro il Parlamento, perché questa è una democrazia parlamentare. La Costituzione non si difende soltanto per motivi strumentali, quando fa comodo, ma la Costituzione si difende sempre. Sempre! *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU

Non intendiamo rinunciare a nulla, non intendiamo rinunciare a quello che vogliamo dire, non intendiamo rinunciare alla discussione parlamentare, alla discussione sulla fiducia, perché finché avremo voce noi ci faremo sentire e non potremo più sopportare soprusi. L'ho detto ai Capigruppo. Presidente, io ho combattuto davanti a tutti i soprusi compiuti in quest'Aula e continuerò a farlo,

Senatrice De Petris, vorrei soltanto rappresentarle che, avendo il Governo ormai posto la fiducia sul maxiemendamento, come lei sa, il maxiemendamento ormai non può più tornare in Commissione. Questo è soltanto per una risposta ad una richiesta cambiato. PRESIDENTE. Mi sembra che ci sia soltanto la proposta della senatrice Bernini, che ha chiesto di spostare la dichiarazione di voto e la votazione finale a domenica.

Senatori Questori... Senatrice Malpezzi, torni al suo posto.

semplice manifestazione di consegna di pagine che per noi non hanno valore *(Commenti dal Gruppo M5S)*, perché non abbiamo avuto la possibilità di leggerle e di analizzarle, il questore Bottici, al posto di calmare gli animi, qualora ce ne fosse stato bisogno, si è permessa di mettermi le mani addosso. *(Vivaci commenti

PRESIDENTE. Siccome sono abituata a verificare tutte le posizioni, se c'è stato qualche atteggiamento offensivo, questo sarà verificato.

Vede, signor Presidente, noi qualche ora fa abbiamo segnalato già alla Presidenza che la senatrice Bottici, nonché Questore del Senato, si era permessa, in un suo intervento, di offendere i senatori del Partito Democratico. Lei ha ritenuto di non fare niente. Lei ha ritenuto che fosse giusto che un Questore del Senato potesse offendere i suoi colleghi. Oggi

il conflitto tra maggioranza e opposizione, certamente dovuto ai tempi con cui la manovra è arrivata, ma ancora più al mancato confronto tra maggioranza e opposizione, prima in Commissione e oggi in quest'Aula. Il confronto, però, non è stato possibile evitarlo con la Commissione europea e la mannaia europea è caduta pesantemente sulla nostra manovra, la manovra di uno dei Paesi fondatori. L'Italia è stata sottoposta a una pessima figura e ha pagato in termini di credibilità, ma anche di perdita del valore del risparmio dei cittadini e delle imprese. Presidente, continuo a parlare, ma penso di parlare a me stesso perché l'Assemblea è al di fuori di ogni controllo e ciò mi dispiace, con piacere, apprezzo che sia presente il ministro Tria e ringrazio i Sottosegretari presenti. Mi dispiace però che non ci siano gli artefici principali di questa manovra che sono i due Vice *Premier*. la loro presenza, ma non perché ascoltassero quello che dico, ma per il rispetto che devono al Parlamento e il rispetto parte dalla testa,

ma non si è potuto evitare il confronto con la Comunità europea, con l'Unione europea; un confronto che è avvenuto facendo precedere in tutti gli organi di stampa il fatto che fosse uno degli

Gruppo FI-BP)*, nell'evitare il confronto diretto tra maggioranza e opposizione sulla legge più importante che regola la vita di tutta la nostra comunità. Ciò non può che dispiacermi e mi dispiace anche quale componente della Commissione lavoro, perché la manovra incide pesantemente sui lavori della nostra Commissione. Ci riferiamo al reddito di cittadinanza, così come a Quota 100 e, perché no, anche al *turnover* nella pubblica amministrazione, che ha effetti diretti per quanto riguarda i dipendenti pubblici, ma anche per chi ogni giorno si confronta con la pubblica amministrazione. Tre grandi temi, affrontati solo parzialmente nella manovra, dove manca ancora il dettaglio normativo. Tre grandi temi che vanno misurati con attenzione e tenuti fuori da una facile propaganda. Sì, da una facile propaganda. Essi riguardano infatti la vita la vita delle persone, il loro reddito, la loro capacità di lottare in una società sempre più esclusiva nel senso letterale e cioè una società che esclude i più deboli. Invece voi: fatto, fatto, fatto! Non può essere questa la risposta, specie quando c'è qualcuno che non riuscirà a passare un Natale felice. Gli italiani però non sono stupidi questo è il vostro difetto; avete peccato anche di presunzione - e stanno capendo che la saggezza, non quella dei capelli bianchi come i miei, ma quella di chi ha studiato, di chi ha costruito qualcosa, di chi lavora, dei pensionati, forse sta tornando di moda. L'onestà, signori del Governo, è un prerequisito per chi fa politica. Poi però bisogna riuscire a comprendere che ogni decisione politica ha effetti sulla vita quotidiana di tutte le persone della nostra Repubblica. Quindi la valutazione della manovra, attraverso le votazioni delle proposte emendative, non sarebbe stato un esercizio inutile, anche perché le modifiche ci sono comunque state e sono state pesantissime, scritte prima dalla burocrazia nostrana - anche lei, ministro Tria, ha collaborato a riscrivere la manovra - e poi dall'euro burocrazia;

Anche se ora subiscono uno slittamento nel tempo per ragioni di copertura finanziaria, la pericolosità rimane per gli anni successivi al 2019, tanto che ci hanno chiesto di fare delle coperture straordinarie, fino a quasi 29 miliardi (non so come farete la manovra dell'anno prossimo, se ancora ci sarete e mi auguro francamente di no), attraverso l'aumento dell'IVA fino al 26,5 per cento. Avete capito cosa significa per i nostri lavoratori, per i nostri cittadini e per le imprese un aumento dell'IVA? Forse non ve ne siete resi conto, ma rimango sul tema del lavoro. 5 Stelle, dovete ricordarvi che il reddito di cittadinanza è attuato nei Paesi dove c'è piena occupazione, c'è piena occupazione, che consente di avere contributi tali da poter sostenere le spese per quei pochi lavoratori che lasciano il mondo del lavoro o che sono In Italia la questione è totalmente diversa perché un terzo dei nostri giovani non lavora. Come fate a promettere un reddito di cittadinanza con i fondi che non avete e che vi ha tagliato ulteriormente l'Unione europea? Siete dei folli. State incitando alla rivoluzione il popolo promettendo cose che non potete mantenere. Questa è la grave accusa che vi faccio.

mi rivolgo al Ministro. Questa manovra fantomatica, riveduta, corretta più volte e non sappiamo se prevalente nelle tinte tra il giallo e il verde sono sicuro che non accontenterà nessuno. Non accontenta voi - ma poco male

Signor Presidente, signor Ministro dell'economia, onorevoli colleghi, il fatto che si siano registrate le sceneggiate che abbiamo visto in questa giornata non può impedirci una riflessione di natura economica sulla legge di bilancio. Altri colleghi del Partito Democratico - che ringrazio per il lavoro svolto in queste settimane e in questi giorni - interverranno per stigmatizzare stigmatizzare l'unicità della procedura che si è seguita. Io mi limito a dire, rivolgendomi per sua tramite, signor Presidente, in particolar modo al Ministro dell'economia, che vi era grande interesse nel mondo per la prima manovra del Governo populista italiano. Il Presidente degli Stati Uniti la settimana scorsa ha discusso e litigato con il Presidente della Federal Reserve*.* Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping ha tenuto un discorso straordinario nel 40° anniversario del grande discorso di Deng Xiaoping. L'economia rallenta a livello mondiale dappertutto. Paesi molto diversi dell'Unione europea come la Francia e l'Ungheria vedono in questo momento manifestazioni di piazza complicate da affrontare

di bilancio è il balcone di Palazzo Chigi, che si apre per la prima volta dal 1982. Allora l'Italia aveva vinto i mondiali. Il Presidente del Consiglio era Giovanni Spadolini. Vi si affaccia il capo del primo partito italiano, nonché Vice *Premier* e Ministro del lavoro,

La stampa italiana ha considerato il riferimento al balcone come un riferimento legato al ventennio fascista. Sicuramente nella storia italiana tanti sono i balconi: chi di noi è più romantico può pensare a Giulietta e Romeo, anche se l'immagine di Casalino e Di Maio non fa lo stesso effetto. Chi di noi invece conosce un po' di politica economica sa che il balcone evoca per i mercati internazionali - lo sa bene il ministro Tria - l'immagine del peggior populismo: il peronismo,

Tutti i mercati internazionali hanno dipinto Di Maio su quel balcone come un neo-peronista e l'immagine del Paese ne ha risentito in modo drammatico. È iniziata una precipitosa retromarcia, signor Presidente. La manovra del popolo è diventata la retromarcia dei populisti e vorrei che restasse agli atti, qui in Senato,

Voi eravate il cambiamento e adesso siete il vecchio e questa vostra continua battaglia procedurale non toglie la realtà per quella che è. La vostra misura economica, la vostra manovra di bilancio non portano il Paese a crescere, se è vero come è vero che già nei primi sei mesi di Governo il PIL ha rallentato i posti di lavoro hanno iniziato a diminuire. Se è vero come è vero che forse otterrete la fiducia - anzi, sicuramente la otterrete - avete però perso la fiducia delle imprese e dei consumatori, semplicemente con la forza dei vostri proclami in libertà. Questa è la discussione che avremmo dovuto fare. Do atto al senatore Bagnai di aver fatto un bellissimo intervento sull'Europa. Non lo condivido, ma ha fatto un bellissimo intervento per raccontare che cos'è l'Europa secondo lui e come va cambiata. Però, signor Presidente, il Senato è stato testimone del fatto che il populismo e il sovranismo nostrani non soltanto soltanto si sono fatti dettare la legge di bilancio da Bruxelles, ma siamo arrivati al paradosso che abbiamo dovuto rinviare una seduta del Senato di un'ora *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)* perché il Presidente del Consiglio non aveva avuto l'autorizzazione dal Commissario lituano e dal Commissario francese.

Quello che però rimane come punto ineludibile e di tristezza di questa discussione non riguarda i rapporti tra Governo e opposizione. Essi sono storicamente complicati e il Presidente sa meglio di chiunque altro, per la sua esperienza, quante volte in quest'Aula l'opposizione ha lamentato il mancato rispetto dei propri diritti. Ora c'è però una cosa diversa, signor Presidente: per la prima volta nella storia del Senato in discussione non è il rapporto tra il Governo e le opposizioni,

essere messa in discussione non è la nostra funzione di fare opposizione. Può piacere o meno, ma quella è. che è stata messa in discussione, con un emendamento al buio, che neanche voi avete letto, è la vostra funzione di rappresentanti del popolo italiano. Perché? Cosa è successo, signor Presidente? È successa una cosa semplice. È successo - termino ripartendo da quel balcone - che vi considerano bravi per andare ad applaudire la notte quando il Vice Presidente del Consiglio deve dare annunci storici all'umanità e partecipare alla cerimonia corale dell'applauso,

Voi siete il partito di maggioranza del Parlamento in questa legislatura e avete il diritto e il dovere di portare a casa i vostri risultati. voi siete stati trattati da questo Governo come si fa con il pubblico dei *talk show*: capaci di applaudire, non capaci di dire alcunché. Potete ingannare tutti una sola volta; potete ingannare qualcuno per sempre; non potrete ingannare tutti per sempre. E oggi, con oggi, è finito il tempo del Governo dei

Signor Presidente, membri del Governo, gentili colleghi, voglio iniziare il mio intervento con una riflessione sul significato della parola fiducia: «sentimento di attesa ottimistica verso qualcuno o qualcosa». Ognuno di noi esercita l'attività di parlamentare, perché ha ottenuto la fiducia dei cittadini. Dobbiamo quindi dare le risposte a coloro ai quali abbiamo dato ascolto. Ciascuno di noi ha quindi il dovere di trasformare in atti legislativi il mandato popolare. È con profondo rammarico che, da parlamentare neoeletta, di trovarmi davanti a un muro dove le proposte, anche ragionevoli, mie e dei miei colleghi rimbalzano indietro, come quando giochi a *squash*. E questo dimostra che chi fa parte di questo Governo, detto del cambiamento, è diventato sordo come chi lo ha preceduto. Anzi, peggio. Io sono membro della Commissione politiche dell'Unione europea, che, come sapete, si occupa di recepire ogni direttiva o regolamento europeo. Ogni singola cosa che interessa la vita pubblica italiana ormai ci viene dettata da Bruxelles e noi la recepiamo. Laddove non venga recepita correttamente nel nostro ordinamento, viene aperta una procedura di infrazione, da sanare. Ora siamo andati oltre. La Commissione europea, cioè un consesso di non eletti da nessuno, ha letteralmente dettato le nuove norme a un Governo guidato da un Presidente del Consiglio non eletto da nessuno. Il Parlamento è stato completamente esautorato dell'esame della manovra e la democrazia è stata messa in soffitta, alla faccia della Costituzione e dei Trattati europei, che devono rispettare anche la nostra legge fondamentale. A Bruxelles hanno avuto gioco facile. Si sono trovati di fronte a un Governo che ha cambiato il disegno di legge diverse volte e a una maggioranza che palesa sempre più le proprie contraddizioni. La ragione è semplice: ci sono due partiti diversissimi tra loro. uno con un programma zapatista e con proposte surreali che ha voluto inserire nella legge di bilancio, perché aveva tratto il proprio consenso dalle promesse contenute in quei punti programmatici. Dall'altra parte, vi è invece un partito storico, che aveva condiviso un programma elettorale liberale e riformatore con l'intera coalizione del centrodestra. Era evidente che fossero due programmi largamente inconciliabili tra loro. E l'elettorato si era chiaramente distinto. L'unico collante tra i due schieramenti così diversi è stata l'idea, alquanto bislacca, che, facendo ulteriore spesa pubblica, questa avrebbe fatto crescere il prodotto interno lordo e contrastato il debole sviluppo del Paese rispetto agli altri Paesi che adottano l'euro. Si sono però dovuti scontrare col fatto che uno non è più uguale a uno, non solo per i 5 Stelle, ma anche per chi sostiene le teorie keynesiane, perché quelle politiche non hanno nulla di espansivo, ma sono solo di spesa. L'unica cosa che non si è fatta mancare l'Italia finora è una spesa corrente in continua ascesa, non di rado allocata male, spesso inefficiente, a volte utilizzata per sperperi. Invece di agire in maniera prioritaria su questa spesa, per riqualificarla, tagliando sprechi, inefficienza, burocrazia, inefficacia nell'allocazione delle risorse, hanno pensato di moltiplicarla. Purtroppo - o per fortuna - è un gioco che all'Europa non è piaciuto. Questa volta si dovrebbe quasi rendere grazie all'Europa matrigna, che in questo caso si è comportata come una madre saggia e lungimirante, che vuole fare rispettare le regole al proprio figlio un po' discolo.

Le regole sul debito e sul *deficit* servono a questo. Non sono numeri scientificamente inattaccabili, ma, tutto sommato, sono numeri che anche l'Italia ha condiviso, firmando i trattati e i regolamenti. Le eccezioni alla regola inflessibile sulla spesa fatta indebitandosi, che limita il ricorso al *deficit*, ci sono già, cara Italia, ci ha detto l'Europa. Vi accordiamo spazi finanziari in *deficit* per le emergenze degli anni precedenti e per quelle nuove: nuove: per l'emergenza migranti, che seppur attenuata continua; per il dissesto idrogeologico che subisce il vostro Paese; spazi per il ponte Morandi, per la manutenzione delle strade danneggiate e per i ponti sul fiume Po. Ma non venite a parlarci di reddito di cittadinanza e nemmeno di rivedere le regole pensionistiche. Ora noi ci auguriamo che quel 2 per cento di *deficit* venga utilizzato veramente per le urgenze di questo Paese. Tra queste, certamente non c'è il reddito di cittadinanza, sul quale il Governo voleva sprecare 9 miliardi di euro. Ora butterà un miliardo sui centri per l'impiego, che non servono assolutamente a nulla. Il problema del lavoro e della disoccupazione rimarrà, perché è una misura assolutamente inutile. Diverso sarebbe stato aiutare coloro che sono rimasti indietro (e per questo serviva un reddito di dignità, come quello che abbiamo proposto noi). Anche la riforma delle pensioni deve seguire misure che rendano più dinamico ed inclusivo il mercato del lavoro, altrimenti il rischio è di mandare in pensione dei lavoratori, di non avere nessuno che prenderà il loro posto, perché in una fase recessiva o di crescita moderata dell'economia difficilmente le imprese assumeranno nuovi lavoratori. *(Richiami del Presidente).* Concludo. Lasciatemelo dire: due forze politiche che volevano imporre un cambiamento al Paese hanno finito per riproporre misure tradizionali, tagli alle agevolazioni alle imprese, nuove tasse, nuove aliquote, interventi micro settoriali in ogni angolo della manovra. Insomma, una manovra che non ha nulla di nuovo, che perpetua antichi vizi della vecchia politica, aggiungendo una totale indifferenza nei confronti di quei parlamentari che potevano apportare, con la loro esperienza del mondo reale, un contributo effettivo e solido. Ricordiamoci che il nostro lavoro è volto a contribuire al bene comune

Signor Presidente, signori del Governo, la discussione sulla questione di fiducia ci consente di fare considerazioni che vanno oltre la triste pagina che il Governo sta scrivendo in questi giorni con il disegno di legge di bilancio. Mi faccia esprimere, Presidente, la preoccupazione, che trova conferma in quello che è successo anche oggi, per il piglio e il modo con cui entrambe le forze di maggioranza hanno interpretato questi mesi di Governo. Hanno cambiato idea su tutto, fatto altisonanti proclami sull'Europa per poi farsi scrivere la finanziaria. Hanno spiegato agli italiani che mai sarebbero scesi sotto il 2,4 per cento di *deficit* e oggi ci presentano una manovra che prevede il 2. Ma c'è un tratto comune che unifica i due *leader* di Lega e 5 Stelle, su cui si sono mostrati coerenti e coesi dall'inizio, ed è la manifestazione costante di un fastidio crescente verso le regole del confronto democratico, una voglia di delegittimare tutte le istituzioni di garanzia, di mettere in discussione l'autonomia delle agenzie fino alla magistratura. Chi, da questi ambiti, che sono quelli che garantiscono tutti, esprime nel proprio ruolo idee ed opinioni che contrastano con quelle della maggioranza, viene denigrato, delegittimato, invitato a candidarsi. Avete l'idea che chi vince comanda, non che governa nel rispetto degli equilibri istituzionali. C'è un'idea della democrazia più simile a quella di Orban che a quella disegnata dai nostri costituenti. Si attacca la stampa e si vuole rendere la vita più difficile all'informazione. E oggi si fa di più in un passaggio decisivo per il Paese, come quello della legge di bilancio: si scavalca il Parlamento, si impedisce la discussione, si umiliano i rappresentanti dei cittadini, tutti i rappresentanti dei cittadini. Chi vince può fare tutto, anche sfidare il buon senso, come si sta facendo con questa finanziaria. Questo è il messaggio: umiliare il Parlamento Questo messaggio è un messaggio nuovo, è un messaggio preoccupante. Non è mai successo. Avete fatto una manovra che serve a far finta di mantenere le promesse, ma non ci riuscite. In compenso, però, essa rischia di mettere il Paese in ginocchio. Non sappiamo cosa resterà del reddito di cittadinanza. Con meno di un terzo delle risorse che avevate promesso di investire, rischia di essere inutile e ininfluente sulla vita delle persone povere. Leggeremo, quando ci sarà un testo su cui discutere, in cosa si tradurrà il reddito di cittadinanza. Ma di una cosa siamo già certi: non solo non sconfiggerà la povertà, ma non produrrà neanche quella crescita dei consumi che, assurdamente, avevate venduto come un effetto positivo del reddito di cittadinanza. Anzi, questa manovra, che blocca l'indicizzazione delle pensioni, non quelle d'oro, ma le pensioni sopra i 1.300 euro, che vieta il cumulo, che aumenta le tasse, ridurrà i consumi. Anche su quota 100, 100, vedremo il provvedimento, che si sta traducendo in un'operazione che consentirà a qualche migliaio di persone di andare in pensione prima, ancora non si sa quando, con meno soldi e con l'illusione che questo procuri lavoro ai giovani. Mentre ciò che è certo è che in questo provvedimento non ci sarà nulla per i giovani, non ci sarà nulla per garantire pensioni decenti a chi andrà in pensione nei prossimi anni, che non beneficerà di quota 100 e che, col contributivo, rischia di andare in pensione col 40 per cento del reddito di lavoro che percepisce. Forse questa era una priorità. D'altra parte, sarà proprio il futuro dei giovani e del Paese a pagare il prezzo più alto di questa di questa finanziaria, il prezzo più alto alla vostra propaganda e alla campagna elettorale delle forze di maggioranza. L'anno prossimo dovremo sterilizzare non 12 miliardi di clausole di salvaguardia, come dobbiamo fare da anni,

Significa non poter più investire sul futuro di questo Paese. Vuol dire che, alla fine, l'IVA dovrà essere aumentata, se vogliamo continuare a mantenere i servizi essenziali. E saranno i più deboli a pagare. Sarà proprio quel popolo che, secondo voi, doveva scrivere la manovra. Forse è questa l'idea che avete del Governo. Saranno i giovani a pagare, perché non si potrà investire sul futuro, sullo sviluppo, sulla ricerca e sulla formazione. formazione. Ci dite, a giustificazione, che avete trovato un debito pubblico altissimo. Fatemi fare una domanda: non lo sapevate, quando avete spiegato in campagna elettorale che il reddito di cittadinanza, quota 100 e la *flat tax* erano sostenibili, che questo Paese aveva un debito pubblico altissimo? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ci avete spiegato che era solo un problema di volontà politica. Ora sapete che non è così:

Adesso usate il gioco per aumentare le entrate. Dov'è finito l'impegno per cancellare, senza se e senza ma, il gioco d'azzardo? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avete fatto un'inutile legge contro la corruzione e ora consentite di fare affidamenti diretti senza gara per appalti fino fino a 150.000 euro, riattivando lo strumento più efficace che noi avevamo tolto, con cui le mafia e i corrotti hanno derubato per anni i cittadini di questo Paese. Senza contare le altre misure: l'abolizione del Sistri, che garantisce la tracciabilità del trasporto dei rifiuti. In un Paese in cui il trasporto illecito di rifiuti è diventata la regola, si elimina l'unico strumento di tracciabilità Ebbene, state facendo tutto questo dopo averci spiegato che eravate contro la corruzione e per la moralità e che avreste cambiato questo Paese. Lo state cambiando in peggio, anche da questo punto di vista. *(Applausi dal per molto tempo - ma noi lo sapevamo - che i dati macroeconomici positivi che si sono registrati negli scorsi anni non corrispondevano a un miglioramento delle condizioni di vita concrete delle persone. È vero, è stato così, ma oggi che peggiorano dovete essere consapevoli che la vita delle persone peggiorerà di gran lunga e soprattutto peggiorerà la vita dei più deboli. Peggiorerà in pochi mesi. Avete fermato il PIL, avete bruciato miliardi mettendo a repentaglio la nostra credibilità come Paese. Avete fatto scendere la fiducia dei consumatori e delle imprese. Avete contribuito a bloccare ciò che - lo diciamo, perché è così - il *jobs act* aveva avviato, cioè una grande operazione sul mercato del lavoro che ha consentito negli ultimi anni di aumentare l'occupazione nel Paese.

per far sì che le imprese investano sul futuro e che riprendano ad assumere. State facendo tutto questo umiliando in Parlamento; non le minoranze, non l'opposizione, ma il Parlamento. Il collega Bagnai ha disegnato, con la solita narrazione propagandista,

Non voglio replicare (non ne ho neanche il tempo), ma voglio dire una cosa: con questa manovra, caro Bagnai, non ci sarà più Stato sociale, ma ce ne sarà ancora meno. Con questa manovra non ci sarà meno povertà, ce ne sarà di più. Non ci sarà più crescita.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa manovra è già stato detto tutto e il contrario di tutto. Questo non stupisce, visto che rimane fino all'ultimo una manovra fantasma e come tutti i fantasmi inquieta. È dannosa per il Paese ed è una follia arrivare agli ultimi giorni dell'anno con il rischio concreto di entrare in esercizio provvisorio e non mettere i parlamentari, espressione del popolo, in condizioni di poter analizzare e discutere il provvedimento più importante per il Paese. Alle molte incognite generali su questa manovra, si affiancano alcune certezze negative: di legge di bilancio prevede, in quattro anni, l'aumento di 70 miliardi di IVA; non c'è un aumento delle pensioni minime e in più avete penalizzato le pensioni sopra i 1.500 euro lordi, con il blocco delle indicizzazioni, trattando come pensionati d'oro onesti lavoratori in pensione. Il cosiddetto reddito di cittadinanza, la misura tanto sbandierata da parte di questa maggioranza, ha fondi risicati e, se sarà implementata, tra sei mesi, distribuirà risorse irrisorie dimostrandosi per quello che è: un insulto alle persone, una presa in giro per il popolo. Avete veicolato il messaggio errato dell'assistenzialismo e per giunta non darete seguito a quanto promesso. Tra le varie certezze negative, c'è ancora la mancanza di incisività sulla Bolkestein, un taglio ai premi INAIL per le aziende limitatissimo e, sempre sul fronte imprese, la mancanza completa di un intervento strutturale di ampio respiro, che sia utile a supportare in maniera sussidiaria le condizioni utili per creare e dare lavoro. Questa è l'ennesima dimostrazione che a questo Governo manca prima di tutto una visione complessiva di cosa si debba fare per lo sviluppo. Senza crescita delle imprese è recessione. Dove non ci sono politiche di sviluppo, non ci sono ipotesi per il futuro e questa manovra delle promesse mancate declina i suoi difetti in tutti i settori, compreso quello dell'agricoltura. Il sottosegretario Manzato è venuto in Commissione non a smentire quello che tutti abbiamo evidenziato, ovvero che i fondi stanziati sono esigui, ma a dirci che è intenzione del Ministero avviare nel futuro tavoli di confronto con tutti gli operatori delle varie filiere produttive. Siamo ancora una volta nel capitolo delle ipotesi per il futuro. Nessuno nega che un intervento di ascolto e confronto sia utile; però, quando si è al Governo, bisogna governare e non procrastinare continuando a fare annunci da campagna elettorale permanente. Le parole del Sottosegretario in Commissione avevano, poi, evidenziato come sul fronte agricoltura - cito testualmente - «il Governo interviene soprattutto per fronteggiare questioni specifiche o particolari emergenze». Tuttavia, quello che Forza Italia ha detto per prima e per molto tempo su questo fronte, non viene recepito. Con i colleghi diciamo dall'autunno della necessità di intervenire a sostegno delle emergenze e dei danni che coinvolgono l'agricoltura sia dal punto di vista atmosferico che da quello della fauna selvatica. Ora, però, per quanto abbiamo potuto vedere, ci si sarebbe aspettati l'individuazione di risorse; ma, a questo punto, le risorse non ci sono. non ci sono. Questo Governo continua, purtroppo, a compiere scelte al massimo ribasso o sulla pelle degli italiani e non mette in bilancio su queste partite risorse sufficienti. Questo a fronte di produzioni agricole talvolta distrutte, come dicevo, dal maltempo e a danni per milioni di euro. Anche su questo fronte il giudizio non può che essere, dunque, negativo, così come negativo è il giudizio su tutta la partita agricoltura, dove si investe zero, e parliamo di un pilastro dell'economia nazionale di importanza capitale. Un settore che offre opportunità occupazionali, di sviluppo, di crescita, tutte parole che a questo Governo non piacciono. Un settore che non è più soltanto lavoro nei campi, ma che è filiera, agroalimentare, *marketing*, un mondo sul quale si deve investire e al quale questo Governo non offre opportunità. La soluzione dei problemi viene posticipata e nel presente si costruiscono misure fortemente recessive. Sulla concretezza prevalgono i proclami ai quali poi non si riesce a dare seguito. Questa manovra è la cartina di tornasole della compagine governativa, dove sembra prevalere un'anima del poi; l'idea che nulla debba essere fatto: né il sostegno all'agricoltura né le grandi opere, né un intervento strutturale e strategico sulla raccolta e sul riciclo dei rifiuti né l'abbassamento delle imposte dirette, e nemmeno la *flat tax*, la tassa piatta e unica che tanto servirebbe al Paese. In conclusione, Forza Italia non può consentire, e non consentirà, che questa visione nichilista prevalga e continuerà a lavorare contro l'idea di un Paese di assistiti e di decrescita infelice che dice no a tutto. Noi vogliamo un futuro virtuoso e libero, nel quale vengono valorizzate le eccellenze, vengono messe le risorse in chiave sussidiaria dove necessario e viene dato lo spazio che merita al fare, al creare, al produrre. Per voi queste cose sono Per voi queste cose sono lontanissime e questa legge di bilancio lo testimonia. Noi continuiamo a lavorare perché al Paese migliore sia dato lo spazio che merita. signori del Governo, colleghi senatori, un grande scrittore calabrese, uno dei uno dei più grandi scrittori della nostra Regione, Corrado Alvaro, nel secolo scorso soleva dire che la gente di Calabria, i calabresi «vogliono essere parlati». In verità, tutti i popoli desiderano di «essere parlati», ognuno va alla ricerca di una parola, ma in quel momento storico, un momento difficile per il Mezzogiorno d'Italia e per la nostra se mai il Mezzogiorno d'Italia in questi ultimi secoli ha vissuto dei momenti facili, voleva dire che c'erano Governi che avrebbero dovuto parlare in maniera diversa alla gente del Mezzogiorno e alla nostra Regione, alla nostra Regione, alla nostra gente. Probabilmente il voto che il MoVimento 5 Stelle è riuscito a prendere il 4 marzo

di più. Il risultato è che questo Governo è sordo alla gente del Mezzogiorno, perché in questa legge della instabilità è rimasto sordo alle richieste della gente del Mezzogiorno ed è muto rispetto alle istanze e alle richieste che in maniera forte erano uscite dalle urne del Mezzogiorno d'Italia, dai seggi del Mezzogiorno d'Italia. Mezzogiorno d'Italia. Mi riferisco a due o tre questioni specifiche che riguardano il Mezzogiorno e anche la mia Regione. Non ha saputo parlare ai lavoratori precari calabresi. Dietro quella sigla ex LSU ed ex LPU ci sono uomini e donne, lavoratori e lavoratrici ai quali noi, nei passati Governi di centrosinistra, abbiamo dato dignità, uomini e donne che oggi lavorano, avviando il processo di stabilizzazione e mettendo in campo le risorse per la proroga e soprattutto per le deroghe. non li avete ascoltati e che non avete saputo parlargli, avete messo in campo le risorse per mantenerli fino all'ottobre del 2019, assumendo che è possibile stabilizzarli nel corso dei prossimi dieci dieci mesi. Non avete saputo parlare alle Regioni, non avete saputo parlare ai municipi del Mezzogiorno d'Italia e della mia Regione, la Calabria. Ho letto la nota dei senatori calabresi che esultano per i nove milioni di euro dati all'aeroporto di Crotone in tre anni. Omettono di dire, però,

legge di instabilità. Ci sono tante ragioni per le quali noi questa legge non la possiamo votare, ma ce ne sono altre due che vorrei sottolineare. Questa doveva essere la legge di stabilità del cambiamento e invece è la legge di stabilità dello sbandamento e dell'arretramento. Voi con questa gloriosa macchina siete andati a sbattere contro il muro dell'Europa; avete fracassato la macchina di questo Governo e in più avete creato lesioni al Paese che sono pericolosissime per quello che potrà accadere alla nostra economia. È la legge perché voi avete risposto alla richiesta forte dei giovani del Mezzogiorno e della mia Regione, che volevano «essere parlati», con il reddito dell'assistenzialismo e non con il reddito della cittadinanza, perché essere cittadini per un giovane significa avere il posto di lavoro. *(Applausi signor Presidente. Se fosse ancora vivo Corrado Alvaro, vi direbbe che non solo non avete saputo parlare agli uomini e alle donne del Mezzogiorno d'Italia, ma che «non sono stati parlati» perché li avete imbrogliati.

per un senatore di prima nomina come me, ma di lungo percorso politico, è qualcosa di incomprensibile, un quadro di Magritte. Confesso uno spaesamento notevole nel non poter in nessuno modo capire che cosa sta accadendo, che cosa stiamo votando, quali decisioni stiamo prendendo. E non mi sento mi sento minorato in questo, perché sfido molti dei miei colleghi presenti in Aula a dimostrarmi il contrario. Peraltro, colleghi, qualcosa è già successo quando abbiamo votato i fondi per le periferie. che è stato ampiamente discusso e sarà molto meglio di me illustrato dai colleghi, a cominciare dal collega De Bertoldi che ha seguito tutta la

qualcuno mi interpella, e credo capiti a tutti voi. Insomma, non è carino dire: «vediamo che cosa succede»; «vediamo che cosa esce»; «andiamo a leggerlo quando lo vedremo approvato». approvato». Personalmente mi reputo un senatore, un senatore della Repubblica italiana, eletto peraltro in un collegio importante, qual è il capoluogo della mia Regione; ho una altissima considerazione del mio ruolo e - se mi consentite - anche di me stesso. Io non valgo uno. Qualcuno qui dentro pensa che uno vale uno, ma seduti in questo scranno non valiamo uno. *(Applausi Colleghi, ognuno di noi, qualcuno meritatamente e qualcuno immeritatamente - ma questa è la democrazia, evidentemente - non vale uno, ma vale uno per ogni voto uno, ma vale uno per ogni voto che ha registrato; e vale uno per ogni istanza portata avanti dalla sua parte politica. È una cosa seria, una cosa importante. Nelle istituzioni gli strappi, gli strappi, come quelli verificatisi in questi giorni e come quello accaduto oggi, sono ferite che si rimarginano male; sono ferite su cui noi, col precedente, mettiamo il sale. Perché il precedente, nel governo delle istituzioni, è una cosa micidiale e non c'è mai fondo. Al peggio non c'è mai fine, non c'è mai fondo; non si rimbalza mai

non è una storia normale, è una storia che va all'epilogo, è un brutto film, signor Presidente. Io credo, spero e voglio

il decoro di questa istituzione sta dentro ognuno di noi ed è nella responsabilità di ognuno di noi. Affrontare gli atti consapevolmente e sapere che cosa abbiamo votato quando usciamo di qui è il minimo indispensabile per esercitare il nostro ruolo. Grazie, colleghi, e scusate se vi ho intrattenuto più del tempo che meritavo. Signor Presidente, voi penserete che io sia intervenuta e vi abbia intrattenuto sin troppo. È per questo, signor Presidente, che le darò una buona notizia: mi sono privata di tre minuti e interverrò solamente per sette minuti.

sulla filosofia che questa manovra non incarna. Benvenuti, in Parlamento, a una manovra scatola vuota, che non ha una stella polare e non ha un'idea di Paese *(Applausi un insieme di piccoli egoismi personali che presidiano un contratto di Governo che rappresenta solo una spartizione di potere. *(Applausi dal tra due partiti che stanno al Governo, diversi, distinti, distanti e che hanno come unico elemento in comune il contratto di Governo. Noi, che crediamo veramente nella democrazia, noi che crediamo veramente che quando le promesse si fanno bisogna mantenerle, abbiamo un unico contratto valido e validato: il contratto che abbiamo stipulato il 4 marzo con il popolo italiano. E non è solo il nostro contratto; è un contratto di centrodestra, un contratto che non prevede l'assistenzialismo e il parassitismo di Stato a scapito dei poveri pensionati che hanno lavorato una vita per guadagnarsi 1.300 euro al mese, che vengono vampirizzati per dare il reddito di cittadinanza ai "disoccupati". Una categoria peraltro che questa manovra a scatola vuota non definisce; è una norma in bianco. Noi portiamo via - ma ci rendiamo conto? - noi portiamo via a persone che hanno la pensione di 1.300 euro al mese, con cui magari mantengono una famiglia figlio disoccupato, il nipote che va all'università, la moglie che fa il telelavoro perché non trova altro, ecco noi portiamo via a questa categoria di persone, da questi 1.300 euro, il reddito di cittadinanza. Cioè voi state colpendo il cuore pulsante del Paese, state massacrando quello che è rimasto del *welfare* italiano. A vantaggio di chi? Di soggetti non meglio identificati, che saranno titolari non di 780 euro (la famosa promessa, 780 euro per 6 milioni di italiani poveri). No. Volendo questo Governo continuare a sventolare le bandierine sbrindellate dei loro provvedimenti *testimonial*, il reddito di cittadinanza non sarà più di 780 euro, ma sarà di 83 euro

hanno 1.300 euro di pensione ogni mese. È una cosa di un'iniquità straordinaria e noi siamo terribilmente arrabbiati per questo. Non possiamo utilizzare altri aggettivi, siamo arrabbiatissimi, ci vergogniamo

un esimio e autorevole rappresentare di questo Governo, il ministro Di Maio, ha identificato una categoria: fatto. Allora 780 euro che diventano 83 euro al mese: fatto. Reddito di cittadinanza sottratto ai pensionati: fatto. 800 milioni sottratti alle Ferrovie dello Stato e quindi ai treni dei pendolari: fatto.

senatrice Bernini, non metta le mani addosso al povero senatore De Poli...

credo abbia rischiato molto di diventare acquiescenza verso la maggioranza e il Governo. Di fatto si sono lasciate calpestare totalmente le prerogative dell'Istituzione, del Senato e di ciascuno dei senatori presenti. Credo che le cose che sono successe, in questi giorni, in quest'Aula non possano essere rubricate a questione squisitamente formale. Qui è stata, nei fatti, calpestata la dignità dell'Istituzione.

riflessioni che riguardano ciò che voi avete detto in campagna elettorale e ciò che i rappresentanti di Governo hanno detto in campagna elettorale. Potremmo fare la differenza tra la campagna elettorale, l'inizio della discussione sulla manovra e il punto in cui siamo arrivati adesso. Si potrebbero fare tantissimi discorsi, ma credo che le questioni più puntuali siano quelle di merito. Mi permetto di citare tre questioni che sono a mio avviso puntuali nel tratteggiare il profilo di come nel concreto la maggioranza si sia calata nella pelle degli italiani. La prima è la questione dell'editoria; aver soppresso di fatto, in prospettiva del 2022, tutti i fondi che andavano a sostenere tanta piccola editoria locale, tante piccole testate che rappresentavano libertà di pensiero, con quotidiani settimanali sui territori, credo sia un atto che si commenta da solo. Aver posto in calce a quell'emendamento l'impegno a varare con decreto ministeriale una norma, che andrà a finanziare progetti scelti dalla Presidenza del Consiglio, credo sia la cifra del passaggio tra un dato di sostegno all'editoria ad un dato che rappresenta la scelta di coloro a cui si darà una mano. Credo che questo sia un tratto caratterizzante. la cancellazione dello sconto sull'Ires per il terzo settore. Si vanno a colpire enti di assistenza, fondazioni, società di mutuo soccorso, istituzioni di assistenza sociale, enti di assistenza e benevolenza, enti religiosi, istituti autonomi delle case popolari,

La terza questione è relativa all'annuncio del taglio delle pensioni d'oro. Avete detto che avreste tagliato le pensioni d'oro. Leggendo però le tabelle economiche della relazione tecnica, si scopre che alle pensioni d'oro tagliate 140 milioni l'anno, mentre invece alle pensioni che superano i 1.200-1.300 euro, attivandovi sulle indicizzazioni, di fatto tagliate, come dice la relazione tecnica,

per il 2020 e 29 miliardi per il 2021. Lasciate sulle spalle delle future generazioni un peso astronomico che comprometterà qualunque tipo di ragionamento sul futuro. Chiudo con una considerazione. Si Si è sentito di tutto in questa Aula: che sarebbe responsabilità dell'Unione europea e responsabilità di tutti. L'altro giorno, nel suo intervento, il senatore Romeo ha detto che questa manovra non c'entra niente con l'Unione europea e che è una manovra che per la prima volta è scritta in Italia dagli italiani. Ecco io credo che il senatore Romeo avesse perfettamente ragione. L'Unione europea ha sicuramente lavorato perché i saldi, la sostenibilità

Signor Presidente, la cosa che a me più ferisce è che poteva essere veramente un'occasione per scommettere sul futuro, sulle potenzialità di sviluppo del Paese e sui giovani. Invece, è un'occasione persa, giocata totalmente alla caccia di consenso spicciolo con piccole misure, senza la capacità di una visione strategica. Io credo che questo sia il danno più grosso. È una straordinaria occasione persa

vorrei iniziare con un numero: 12.147.000 sono i voti che il centrodestra ha preso alle elezioni del 4 marzo. marzo. Presidente, in questo Senato - lei lo sa meglio di me - ci sono 23 senatori di Forza Italia eletti con il sistema maggioritario e ce ne sono 19 della Lega eletti allo stesso modo. Sono 44 persone che hanno preso i voti da tutti i nostri elettori indistintamente.

Poi ce ne sono altri al Sud, ma non avendo avuto i voti della Lega, che all'epoca era quasi inesistente, sono rimasti a casa o altri sono stati eletti nel sistema proporzionale. In ogni caso, abbiamo combattuto la stessa identica battaglia e i nostri avversari sono quelli che siedono al centro e a sinistra di questo Parlamento. Ciò serve a dire che siamo sicuramente una famiglia politica che ormai da circa venticinque anni lavora per il bene degli italiani. Possiamo pensare di dissolvere tutto questo? No, io credo proprio di no.

Se qualcuno vi ha detto che potevate farlo, secondo me ha sbagliato. È stato grave, anzi, gravissimo, ma non un errore nostro. Siete stati voi a farlo perché avete aderito. In questi mesi dal contratto di Governo ad oggi sono stati smarriti tutti o quasi tutti i principi per i quali abbiamo chiesto il voto ai nostri lettori il 4 marzo. il 4 marzo. L'unica cosa decente è la vicenda sulla Bolkestein, sulla quale abbiamo combattuto anni insieme e forse - visto che c'è il ministro Centinaio - si poteva o si doveva fare di più, ma capisco

Se qualcuno avesse dei dubbi, in ogni caso, ci sono le sceneggiate di queste due settimane e quelle di oggi, tra Commissione e Assemblea, senza aver mai votato un emendamento.

risulta incompleto e frutto di compromessi, che non vanno nella direzione degli interessi degli italiani. Quindi gli italiani si sono tolti ogni dubbio sulla vostra totale incapacità di governare. Veniamo dunque i numeri sono importanti. Ieri mattina il Governo ci ha detto - o meglio, ha tentato di dirci - che per valorizzare il lavoro svolto ha enfatizzato alcune misure, che ha dichiarato essere alcune delle tante contenute in questa manovra, che noi però non conosciamo, visto che non abbiamo avuto neanche il tempo di leggere il maxiemendamento. una riflessione in particolare sugli enti locali. Vi siete arrogati il merito di aver risolto la questione dell'avanzo di amministrazione di poterlo spendere. Ebbene, se non fosse stato per la Corte costituzionale, che attraverso una propria decisione, contro una scelta scellerata di un provvedimento emesso dal Governo di centrosinistra di qualche anno fa, che bloccava la possibilità dei Comuni di spendere ciò che i propri cittadini avevano già pagato con le tasse,

per consentire loro di trattenere l'IMU che viene pagata dalle famiglie e dalle imprese? Non eravamo noi - e quando parlo di noi, mi riferisco a noi di Forza Italia e a voi, colleghi della Lega - che dicevamo che le tasse pagate da un territorio dovessero restare su quel territorio e non entrare nel calderone dello Stato? Non siete voi che state minacciando una crisi di Governo se non vi portano in Consiglio dei ministri l'autorizzazione all'autonomia delle Regioni del Nord?

che vengono drenati, con l'aumento dell'Ires alle associazioni no-profit per i disabili, che passa dal 12 al 24

C'è un documento dell'Unione delle Province italiane che dice che le Province hanno bisogno di 1,5 miliardi di euro per gli investimenti, le strade e gli istituti scolastici e di 280 milioni di euro per la spesa corrente. Conoscete la differenza tra spesa corrente e investimenti? Signor Presidente, concludo, saltando molte delle cose che avrei voluto dire. Mi faccia dire un'ultima cosa sulle pensioni. Per recuperare 2,2 miliardi di euro e contrabbandando il taglio a pensioni d'oro (che sono 24.600 su un totale di 16.100.000 pensionati), voi andate a togliere a coloro i quali percepiscono da 650 a 1.600 euro al mese un pezzo del loro futuro, tagliando fino al 48 per cento l'incremento della loro pensione per l'anno 2019. Questa è una vergogna. *(Applausi dai manovra del cambiamento, noi facciamo bene a votare contro anche senza avere letto il maxiemendamento.

Meritate l'alloro per l'abilità di dire una cosa e, poi, fare esattamente il contrario e di camuffare il tutto con una viscida gelatina di menzogne, una disinvoltura e un'arroganza di cui peraltro è davvero difficile trovare precedenti. Oggi ricorrete al paracadute del voto di fiducia, mascherando una discussione strozzata, mai come questa volta, su un provvedimento - anzi, sul provvedimento - più importante che la nostra Repubblica è chiamata ad adottare e che voi non siete stati in grado di sottoporre all'attenzione delle due Camere, così come avreste dovuto fare fin dallo scorso 20 ottobre. Solo oggi, agli esiti di una discussione finta e di un teatrino, di scuola casaliniana, architettato solo per nascondere la verità i numeri dettati dai burocrati di Bruxelles (quei burocrati così tanto bistrattati in campagna elettorale), prende luce un provvedimento rabberciato, che necessita di essere approvato dalla due Camere in una manciata di giorni e che è pieno zeppo di strafalcioni. Penso alle vicende degli NCC e del demanio, che regaleranno all'Italia solo altre procedure di infrazione, che costeranno altri soldi agli italiani e non risolveranno le aspettative che colpevolmente avete alimentato. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ecco, dunque, il ricorso alla fiducia, quella stessa fiducia che solo qualche mese fa avreste tacciato come golpista e metodo da dittatura. E allora vi chiedo: quella a cui oggi fate ricorso, di grazia, come la chiamate? Come definite la negazione senza precedenti del dibattito nella sessione di bilancio?

urlato, violento e ad oltranza, quello stesso ostruzionismo che nella precedente legislatura ha dato notorietà a gran parte degli esponenti dell'attuale Governo. Avreste certamente occupato i banchi della Presidenza e del Governo e inneggiato alla rivoluzione del popolo. Noi invece no, non lo facciamo. Vorrei fosse chiara la differenza tra voi e noi: noi siamo un'altra cosa per responsabilità, senso delle istituzioni e serietà.

per i presupposti di questa manovra, che qualcuno sostiene - a ragione - avrebbero paradossalmente reso l'esercizio provvisorio il male minore.

Ci presentate la manovra di un re senza più corona né scettro; un disegno di legge di bilancio firmato da sovranisti senza più sovranità, che - paradosso tra i paradossi - non ci sottrae del tutto dal rischio di procedura di infrazione e, dunque, di una possibile nuova austerità. Certo - tengo a precisarlo e mi dispiace che il ministro Tria si sia di nuovo allontanato - eravamo contenti che si fosse evitata, almeno per ora, la procedura di infrazione per *deficit* eccessivo. Non siamo mai stati tifosi dello *spread*, ma favorevoli a tutelare gli interessi del Paese. Siamo, però, arrivati fino a questo punto perché è stato commesso un fiume di errori, che il Governo ha scaricato sul Paese e sulla credibilità dell'Italia, mettendo il Parlamento nelle condizioni, alla Camera, una legge che non era scritta e, al Senato, di dover chiedere invano conto di numeri e cifre che avete ostinatamente nascosto e negato alla discussione. Quella che la vostra spacconeria aveva ironizzato come la letterina di Babbo Natale è diventata la missiva amara che, per vostra mano, la Commissione europea notifica all'Italia *(Applausi

e, in termini politici, una retromarcia mai vista; un'affermazione di subalternità che solo gli occhi della propaganda, anche degli accademici prestati alla propaganda, riescono a non vedere. Domando: non eravate voi gli oratori dei tempi dell'opposizione o, appena pochi mesi fa, in campagna elettorale, coloro che battevano i pugni a Bruxelles? Quegli stessi pugni ora, però, cosa stringono? Forse stringono un pugno di mosche, a danno di un Paese intero, del suo futuro, del suo sistema di imprese, del Mezzogiorno. Il presidente Conte avrebbe dovuto essere qui anche questa sera ad ammettere che vi siete sbagliati a fare i conti sui costi di quota 100 e reddito di cittadinanza, assumendosi la responsabilità, perché tutto ciò è già costato almeno un miliardo e mezzo di euro, e questa cifra è stata pagata per intero dagli italiani, dalle imprese e dai risparmiatori. Certo, dall'avvocato del popolo ci saremmo aspettati ben altro: un soprassalto di dignità, un esercizio di verità. E invece no: ha continuato anche lui, imperterrito, la retorica del Governo del cambiamento, della campagna elettorale perenne, tutto sulla pelle degli italiani. Così la riscrittura fatta a Bruxelles ci consegna una manovra recessiva, in cui non ci sono misure per la crescita, né per gli investimenti, che penalizza le imprese, mortifica il Sud con pesantissimi tagli ai cofinanziamenti sui fondi Regionali, blocca il *turnover* nella pubblica amministrazione; una manovra che smaschera la propaganda di un reddito di cittadinanza e quota 100 dei quali resta poco più del titolo e la barzelletta incerta sui tempi di attivazione. Ecco in cosa si materializzano gli 11 miliardi di tagli nel 2019. Ripeto quanto ho già detto ieri: urla vendetta la riduzione di almeno 700 milioni di euro di fondi per le Regioni, già stanziati per cofinanziare i fondi strutturali europei. Altro che messa in sicurezza del Paese! Come urla vendetta il taglio di 800 milioni di euro dalla riprogrammazione del fondo di sviluppo e coesione. PD e del senatore Vitali)*. Ma urla vendetta anche il taglio di 850 milioni alla rimodulazione dei fondi di cofinanziamento nazionale: un vero e proprio martirio, che peserà almeno per due miliardi e mezzo sulla testa delle imprese. Ma avete fatto ancora peggio: con una scellerata cocciutaggine, invece di concentrare risorse per accompagnare i timidi ma chiari segnali di crescita registrati per più trimestri e fino all'avvio di questo Governo, cosa fate? Escogitate un taglio di 410 milioni di euro per colpire direttamente le agevolazioni alle imprese, attraverso i quali limate il credito d'imposta IRAP e azzerate totalmente - dico, azzerate quello per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Tagliate i fondi di agevolazione Ires e poi - giusto per farsi del male fino in fondo - vi producete in un taglio per ridurre anche lo stanziamento di risorse per il capitale immateriale.

di voler aumentare la domanda interna, che era alla base della vostra stima eccessiva di crescita più alta del PIL. Vi ricordate tutto questo teatrino? E poi che fate?

entra nelle tasche degli italiani. L'IVA taglia le banconote nel portafoglio: altro che chiacchiere. Componenti del Governo, davvero pensate di continuare a prendere in giro gli italiani? È vergognoso che non proviate un senso di vergogna per quello che state facendo. Per colpa Per colpa vostra quest'Aula questa volta voterà una fiducia al buio, su un testo partorito di notte e votato di notte;

«Si avanza nel buio a tentoni fin dove, invano prevista, si apre sotto i piedi la botola», scriverebbe un poeta. Io spero che quella botola non si apra del tutto, che quella voragine che state scavando sotto i nostri piedi non ingoi per sempre la speranza di questo Paese.

«il Governo non si azzardi a presentare al Senato il maxiemendamento sulla legge di bilancio per farlo poi passare in fretta e furia con l'ennesimo voto di fiducia e, infine, farlo

che priva il Parlamento delle sue legittime prerogative. Abbiamo già avvertito i Presidenti di Camera e Senato e i Presidenti della Commissione bilancio. Se non ci faranno discutere il testo nel merito, li faremo rimanere qui

all'eversione, al *golpe*, alla dittatura. Avete assalito, furiosi, i banchi del Governo. Avevate promesso di aprire il Parlamento ai cittadini e l'avete trasformato in un guscio vuoto, mortificando le istituzioni di questo Paese. Avete ridotto il luogo sacro della democrazia all'irrilevanza. all'irrilevanza. Lo avete umiliato e, agendo in questo modo, avete umiliato i cittadini elettori che ci hanno dato il mandato. Li avete umiliati voi stessi. State attentando alla Costituzione della Repubblica. State stravolgendo anche il principio della distribuzione dell'equilibrio tra i poteri dello Stato. Oggi l'abbiamo visto plasticamente e lo hanno visto anche i cittadini da casa. Siete turisti della democrazia, perché non la praticate. Siete pericolosi. Siamo stati eletti per leggerle la manovra, per portare il nostro contributo, per valutarla con coscienza e nell'interesse degli italiani, anche di quelli che hanno eletto noi, perché non hanno eletto solamente voi. Fatevene una ragione: hanno eletto anche noi. Ce lo state impedendo. Ce lo avete impedito e avete messo il bavaglio al Parlamento. La collega Rauti ieri ricordava che siamo qui ad aspettare Godot, come in una sorta di commedia dell'assurdo. E, per ricalcare le citazioni letterarie, vorrei dare un suggerimento di lettura o di rilettura, ammesso che qualcun altro lo abbia letto: «Cecità» di Saramago, e non perché qualcuno possa pensare che stiamo facendo una manovra al buio, per quanto sia vero, ma perché perché la cecità è l'indifferenza con cui voi, colleghi parlamentari, accettate passivamente questo strappo che lede anche il vostro ruolo, perché non avete contribuito neppure voi alla stesura

Entriamo però nel merito, perché voglio dirvi perché vi diciamo no. La manovra doveva essere lo specchio del vostro contratto, costruito sugli *slogan* della vostra campagna elettorale: reddito di cittadinanza da una parte, azzeramento della Fornero dall'altra. La maggioranza - e in questo noi crediamo - ha l'onere Non siete stati, però, in grado neppure di garantire, in minima parte, alcune delle promesse - per noi sbagliate - che avete fatto in campagna elettorale. Non c'è il reddito come lo avevate raccontato e non c'è l'abolizione della Fornero. Piuttosto, c'è un furto ai pensionati a 1.300 euro e il furto delle illusioni di chi si aspettava 780 euro e ne riceverà meno di 100,

di quelli che mi stanno più a cuore, occupandomi da una vita di futuro, essendo un insegnante. Di futuro in questa manovra non c'è nulla, perché non avete previsto nulla per scuola, cultura, università, ricerca, innovazione digitale e formazione, anche se avete il coraggio di scrivere sulle veline di regime, che mandate in giro sui *social*, in cui siete fortissimi, che avete fatto il tempo pieno nelle scuole. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma davvero avete il coraggio di dire che con l'assunzione di 2.000 avete fatto il tempo pieno nelle scuole e avete risolto il problema? Fermo restando che con il decreto disoccupazione del vostro ministro Di Maio di insegnanti ne avete licenziati in tronco 5.000, il saldo è comunque negativo; su questo potete davvero mettere la spunta. Ne servirebbero 41.000 di docenti per fare il vero tempo pieno. Eppure, in campagna elettorale avevate parlato di investimenti per miliardi di euro sulla scuola: ve lo ricordate? Che credibilità avete? Su una manovra da 27 miliardi avete speso per la scuola 25 milioni. Avete cancellato la formazione iniziale degli insegnanti, perché non vi interessa che siano preparati, ma vi interessa fare cassa. Così 12 milioni li avete messi da parte. D'altra parte cosa ha detto il ministro Bussetti? La scuola faccia con quello che ha. Ora metteteci la faccia di fronte a questa affermazione; andate nelle scuole a dire che devono farcela con quello che hanno. Voi non credete nel capitale umano dei nostri ragazzi, quelli che invece di mandare a lavorare volete tenere inchiodati ai sussidi o al divano, come ha detto Salvini. Dobbiamo invece - noi che ci crediamo - investire sulle nuove generazioni. voi niente di niente: di scuola, formazione e università. Nell'era del cambiamento si parla solo del presepe natalizio, dei compiti da non fare durante le vacanze, degli indegni regolamenti per escludere i bambini dalle mense scolastiche, delle telecamere fuori dai plessi o cani antidroga: bellissima visione che avete della scuola. Vi diciamo no, perché a voi dei giovani non interessa nulla. Voi, nel secondo Paese più vecchio al mondo, dove la disoccupazione dove la disoccupazione giovanile è sempre troppo alta e dove i risultati degli apprendimenti certificano ritardi da colmare, non mettete un euro sul futuro dei giovani, ma fate ciò che di più triste potrà esserci: scommettere sul loro fallimento per poi dargli chiaramente 83 euro

Cambiare significa dare opportunità, costruire il futuro, valorizzare il nostro straordinario patrimonio. Ma voi cosa fate? Tagliate anche sulla cultura che con voi è destinata a una lenta e inesorabile estinzione: tagli e riduzioni colpiscono indiscriminatamente librerie, case editrici, sale cinematografiche, musei autonomi e il *bonus* cultura per i diciottenni. la serie di pesanti sforbiciate lasceranno il segno inequivocabile delle vostre scelte. Ma voi vi nutrite del degrado, che è la benzina del vostro consenso, e allora perché dovreste combatterlo? Oltre ad aver mortificato la cultura, avete minacciato e attaccato la libertà di stampa e i giornalisti, consapevoli che la libertà di stampa è uno dei principi fondamentali della vita democratica. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma per voi la democrazia è l'inutile orpello, il fastidio, l'ostacolo tra voi e il popolo. voi e il popolo. Ve lo ha insegnato Casaleggio: vi ha detto che il Parlamento è inutile, non vi serve, non ci serve. Vi siete vantati di aver messo 60 milioni sull'università e la ricerca. Sapete quanto valgono nei 27 miliardi? Valgono solo l'aumento di 40 milioni del Fondo di finanziamento ordinario, di cui il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico senza vergogna si vanta, è irrisorio rispetto alle risorse

Bloccate le assunzioni a tempo indeterminato anche nelle università. E questo colpisce quella fascia anagrafica tra i trenta e i trentacinque anni preparata, competente e contendibile a livello internazionale, che rischiamo di perdere.

2017. Nulla è ancora arrivato da questo Governo. Voi, che dovevate abolire la povertà, avete abolito il futuro e la speranza. Il Paese - statene certi - non vi perdonerà.

quello che sta accadendo con questa manovra è qualcosa che non ha precedenti nella storia della Repubblica: si deve tornare forse addirittura ai tempi dell'antica Roma - quando Caligola nominò senatore il proprio cavallo per rintracciare una tale delegittimazione del Parlamento, o ancora al Venezuela di Chavez per vedere una manipolazione dell'opinione pubblica, una demagogia populista che si prende gioco dei cittadini, quale è la strategia messa in atto da questo Governo. Finché quest'Assemblea, almeno sulla carta, continuerà a contare qualcosa, abbiamo il dovere di denunciare lo scempio che si sta compiendo alle spalle degli italiani. Avete alzato il livello dello scontro con l'Europa, difendendo misure insostenibili, come il reddito di cittadinanza e quota 100. Avete bruciato miliardi, fatto impennare lo *spread*. Avete scritto una manovra senza investimenti, ma piena solo di *spot* elettorali. Avete alterato le stime di crescita. Avete portato l'Italia sull'orlo della procedura di infrazione. Avete ingaggiato una lotta di principio, per poi - dopo che per mesi vi avevano invitati a fare marcia indietro, dopo aver parlato di sovranismo, Italia agli italiani, invocato poteri forti che remano contro il Paese alzare le mani e consegnare il destino del popolo italiano a Bruxelles, che ha corretto il compito dell'alunno somaro, lasciando dentro qualche misura *spot* degna al massimo di un manifesto elettorale. Reddito di cittadinanza, anziché misure che incentivassero l'occupazione: un provvedimento che aumenterà semplicemente il lavoro nero e peserà sulle casse dello Stato. La *flat tax*? Dimenticata, sostituita da un banale allargamento del regime forfettario. Vi svelerò un segreto: defiscalizzare crea occupazione.

Siete riusciti in qualcosa di incredibile: avete tradito gli imprenditori, avete tradito la classe media e persino chi vive sotto la soglia di povertà. Vogliamo poi parlare delle pensioni? Avete detto che avreste aiutato i pensionati. Avete fatto becera propaganda sulle pensioni d'oro, ma poi avete bloccato le indicizzazioni di quelle sopra ai 1.500 euro. soprattutto, avete introdotto quota 100, ma nella manovra avete però bloccato le assunzioni nella pubblica amministrazione per tutto il 2019. Avete addirittura introdotto un blocco delle assunzioni nelle università, lasciando a piedi i giovani ricercatori che tanto fanno per questo Paese. Volete spiegare come saranno sostituiti i lavoratori che andranno in pensione, se bloccate nei fatti e al di là delle parole le assunzioni, in settori poi come le università, che sono la linfa in cui cresce e si forma la classe dirigente del domani? Vogliamo poi ricordare come avete attaccato la stampa - come è stato detto poco fa - punita con i tagli all'editoria, colpevole di raccontare la verità ai cittadini che avete tentato di prendere in giro, raccontando di un *deficit* al 2,04 anziché al 2,4, sperando che non si accorgessero di quello zero di troppo? una trovata di cui, a quanto apprendo proprio dalla stampa, il portavoce del *premier* Conte, Casalino, si vanta ancora; becera propaganda, che dal *web*, in cui diffondente quotidianamente *fake news*, avete trasportato nelle stanze delle istituzioni. propaganda non l'avete risparmiata neppure ai terremotati, promettendo loro di ridurre del 40 per cento i tributi dovuti - così come fece il Governo Berlusconi in occasione del sisma di L'Aquila

creando una disparità di trattamento tra i cittadini di L'Aquila e quelli, ad esempio, di altre Regioni e di altre Province del Centro Italia. E non è giusto. E adesso ci chiedete non solo di approvare la vostra manovra, ma anche di dare la fiducia a questo Governo; un Governo che, fino ad ora, ha prodotto solo misure devastanti per il Paese, a partire dal decreto dignità, che ha contribuito a diminuire ancora i posti di lavoro e a mettere in ginocchio le imprese, già prostrate, con la follia delle chiusure domenicali. Per continuare poi con la follia assoluta del decreto che voi avete chiamato spazzacorrotti, un'altra misura degna del Venezuela di Maduro che tanto piace al MoVimento 5 Stelle. Vi suggerirei, in merito, di leggere il rapporto Greco rapporto Greco sull'Italia: il gruppo di Stati contro la corruzione ci chiede di intervenire sui regolamenti interni dei Gruppi in Parlamento. Un accenno, forse, a quei Gruppi che violando la Costituzione, introducono l'obbligo di mandato imperativo, comminando penali-truffa a quei parlamentari in dissenso con il proprio partito? Il vostro provvedimento, bocciato anche dal Consiglio superiore della magistratura, al contrario, non interviene su tutto ciò, limitandosi a trasformare gli uffici pubblici in luoghi di spia, invidia e terrore, abolendo la prescrizione e introducendo processi senza fine, che violano le norme sulla ragionevole durata del processo contenute nell'articolo 6 della CEDU e nell'articolo 111 della nostra Costituzione, e che se ne fregano del principio sancito nella Carta di una pena che deve invece tendere alla rieducazione del condannato. Voi che parlate di taglio agli sprechi, avete idea del denaro che lo Stato dovrà sborsare, in base alla legge Pinto, per risarcire le vittime di processi troppo lunghi? No, non credo che abbiate idea di tutto ciò. Per tutto questo e per molto altro, voteremo no a questa manovra, né daremo la fiducia a questo Governo.

costruttivo ma anche combattuto, e per spirito di opposizione patriottica, voglio entrare in un merito specifico, anzi in due. Mi riferisco - vorrei davvero l'attenzione del Governo al comma 326 in cui, nell'ambito delle disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, con legge di riferimento, si parla di indennizzo corrisposto in favore del coniuge superstite. Vi prego di fare una specifica

semplice ma gravissima dimenticanza, andremo a legittimare casi che la cronaca ha restituito, paradossali ma che si sono verificati, di autori di omicidi che, rimessi in libertà, hanno potuto godere della reversibilità della pensione

C'è un altro punto di merito sul quale voglio e sento di dover intervenire in quest'Aula. Mi riferisco al comma 255 relativamente all'incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica per un totale di 5 milioni. Sicuramente è bene incrementare il Fondo, ma lasciate che io dica, senza voler polemizzare su questa materia, che non si risparmia però sugli orfani di femminicidio. Voi stessi avevate immaginato un incremento di 12 milioni di euro, mentre la misura ne prevede 5. Voglio anche dire che in Commissione bilancio alla Camera avete bocciato un emendamento che proponeva 12 milioni di incremento.

lo avete fatto vostro, ma avete ritoccato al ribasso drammaticamente le cifre, perché siete scesi da 12 milioni 5 milioni. La richiesta era di 2 milioni per le borse di studio e le attività di formazione (ed è rimasta), e ancora di 10 milioni per quelle famiglie affidatarie di orfani di femminicidio, e cioè per quei parenti, nella maggior parte dei casi nonni,

gli autori dell'omicidio sono i padri degli stessi bambini. Alle famiglie di quei bambini - ricordo che non sono numeri ma orfani di femminicidio, bambini a cui è stata uccisa la madre

se avete trovato i fondi per i professionisti del divano, se avete investito tanto e urlato sul reddito di cittadinanza, qualche soldo in più per gli orfani di femminicidio dovevate e potevate trovarlo. Poiché la matematica non è un'opinione - e la politica deve anche ragionare in termini di matematica - e siccome gli orfani di femminicidio sono meno di 2.000, se dividete le somme che avete stanziato per il numero degli orfani, capirete che si tratta veramente e vergognosamente di pochi spicci. Non si risparmia sugli orfani di femminicidio, non si risparmia sui bambini, non si finanziano i divanisti a danno degli orfani di femminicidio! *(Applausi

3.100 donne uccise lasciando figli dal 2000 a oggi. E allora a queste vittime collaterali il Governo deve dare, con senso di responsabilità, maggiore sostegno. A quei 3 miliardi stanziati dal precedente

di tutti e, se posso permettermi, le do la mia personale solidarietà.

sul vergognoso *iter* di questa manovra in realtà è stato detto tutto da tanti, forse tantissimi. Finalmente pare che la manovra sia stata avvistata e forse qualcuno l'ha letta.

signor Presidente, un intervento di sola e forse inutile testimonianza, perché tanto non lo ascolteranno e non lo ascolterete. È come se il passaggio al Senato di questo maxiemendamento, deciso da pochi, anzi direi pochissimi, fosse solo una fastidiosa formalità.

per palese e manifesta incompetenza e malafede. C'è chi, invece, pensa di poter ancora giocare con il bilancio dello Stato come con il pallottoliere, giocare con i risparmi degli italiani a suon di *post* e dichiarazioni come fuochi d'artificio; e magari ci ridono anche sopra con arroganza. Mai vista un'accozzaglia così. TAV sì, anzi no, forse la sospendiamo. I soldi ci sono, 9 miliardi, 18, anzi sono 37, cinquina e tombola. Spezzeremo le reni all'Europa, viva l'Europa, più tardi telefoniamo all'Europa, chi se ne frega dell'Europa, stasera a cena dall'Europa. E ancora: no euro, viva l'euro. L'Ilva la chiudo, forse la riapro, grande successo per l'Ilva. Fornero no, Fornero forse, Fornero forse un po'. 2,4 sì, 2,4 forse, vabbè, facciamo 2,04. Per i bambini non servono i vaccini; per i trasporti non servono le infrastrutture; per i disoccupati non serve creare lavoro; per fare il Ministro non è necessaria la competenza. Ai più volenterosi dei Ministri 5 Stelle proporrei tre tracce. Storia contemporanea: chi era il commissario Calabresi? Geografia: esiste il *tunnel* al Brennero? Economia: come si calcola il PIL?

I cittadini vanno informati a 370 gradi? Fatto. Portati colazione e caffè a Juncker: fatto. Bugie sul *deficit* dal 2,4 al 2,04: fatto.

truffa sul reddito di cittadinanza, da 780 a 83 euro mensili; niente pagamento dei debiti della pubblica amministrazione; blocco dell'indicizzazione delle pensioni da 1.500 euro; via la *flat tax*, IVA in due cancellati gli investimenti per ferrovie e cantieri; Sud abbandonato; ridotto credito imposta; militari tappabuchi, e una collega ieri ha detto che si è passati dalle truppe d'assalto delle assunzioni pubbliche; massacrato il risparmio degli italiani e BTP invenduti; ecotassa non solo sui SUV; tagli e bavagli all'editoria; Italia in recessione: fatto? Fatto! Per dare un'illusione di reddito di cittadinanza ammazzate la classe media; per finanziare il vostro clientelismo elettorale ammazzate tutti gli italiani. Voi, i nuovi, i diversi, quelli che non erano casta, quelli che hanno sbraitato per anni di rispetto del Parlamento, di competenza, meritocrazia e preparazione, avete fatto peggio di Monti e Renzi Apoteosi del fancazzismo eletto a filosofia sociale; il vostro credo è la filosofia del fallimento, il credo degli ignoranti, il vangelo dell'invidia; la vostra caratteristica intrinseca è la condivisione della povertà. Quindi, votatevela questa manovra scritta dagli altri e poi, dopo l'approvazione della manovra contro il popolo, esultate platealmente e potrete dire: fatto! La credibilità, cari colleghi 5 Stelle, è come la verginità: difficile da mantenere, facile da perdere, impossibile da recuperare, e voi l'avete persa. La fiducia: chi più la mette meno la merita e voi non la meritate.

i ritardi importanti che abbiamo registrato qui in Senato sui tempi, ma anche le critiche sulle modalità di approvazione della manovra economica dello Stato sono già stati oggetto, in precedenza e anche questa sera, degli interventi di tante colleghe e colleghi che sono intervenuti. Sicuramente le cause sono da individuare in tutti i passaggi politici e tecnici di una nuova manovra economica portata avanti nei mesi scorsi in modo molto muscolare ed intransigente. Sono state fatte delle scelte sicuramente di rottura, come il reddito di cittadinanza e la quota 100 sulle pensioni, che personalmente vorrei riservarmi di valutare fra qualche mese per vedere le reali ricadute sui cittadini. È quindi comprensibile che tutto ciò abbia portato a dei rallentamenti, soprattutto legati ai passaggi nelle interlocuzioni nei rapporti con l'Unione europea. Ritengo tuttavia che la causa principale del ragguardevole ritardo e dell'incertezza generale degli ultimi giorni sia da individuare nei rapporti fra due partiti di maggioranza. Forse ora i nodi vengono al pettine e i tagli previsti per rimodulare la manovra sono stati l'oggetto del lungo contendere. Un tema - ad esempio - è quello dell'autonomia delle due grandi Regioni del Nord, il Veneto e la Lombardia, e relativi oneri finanziari ritengo sia stato uno dei nodi da sciogliere, argomento che peraltro noi autonomisti seguiamo con attenzione. Tuttavia, a mia volta, devo sottolineare che è stata negata la possibilità a tutti i senatori di poter contribuire al miglioramento di questa manovra. Non vi sono stati alcun voto in queste settimane, nessuna discussione di merito su alcun argomento: nulla di nulla. Il Parlamento della Repubblica è stato - mi duole dirlo - retrocesso a mero passaggio formale e questo è gravissimo. Detto questo, vorrei entrare nel merito del presente disegno di legge di bilancio. La prima cosa che mi sento di sottolineare come componente di un Gruppo Parlamentare che rappresenta le autonomie alpine e, quindi, la montagna, è la scarsa considerazione delle politiche ad essa legate. È noto a tutti come l'ambiente montano sia meraviglioso, ma per certi versi anche molto impegnativo,

ad esempio, dai professionisti del turismo, dai lavoratori di alta montagna e dagli agricoltori, per introdurre dei miglioramenti che andassero a qualificare meglio la manovra. Parlo di sgravi fiscali per imprese turistiche, come quelli relative all'assunzione del personale a tempo indeterminato e stagionale, beni strumentali e canone Rai. Parlo anche del rilancio degli stabilimenti termali attraverso accordi transfrontalieri per rilanciare il turismo della salute ad esso collegato.

più di 4 milioni di euro per finanziare il sostegno all'attività agropascolare di alta montagna. La nostra è un'agricoltura eroica che merita un'attenzione particolare e che però con grande dispiacere non trovo nella manovra. Negli interventi sulla previdenza non vi è poi traccia della volontà di riconoscere il carattere usurante delle attività dei lavoratori della montagna: guide alpine, guardaparco, addetti agli impianti di risalita e maestri di sci, tanto per citarne alcune, che proprio per l'esposizione costante a climi rigidi meriterebbero una considerazione dal punto di vista pensionistico. Non c'è neppure traccia della possibilità da me rilevata di una esenzione dai pedaggi autostradali per Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile nelle loro funzioni di soccorso. Nelle attività produttive e in quello delle energie rinnovabili spiace ancora constatare la scarsa attenzione da parte del Governo verso la produzione idroelettrica, l'energia pulita che rappresenta uno dei gioielli della nostra realtà montana. Spero vivamente in un cambio di atteggiamento della maggioranza nei confronti di un settore così strategico per tutte le Regioni dell'arco alpino e so che in questi giorni c'è un braccio di ferro con le Regioni e il Governo su questo tema. Abbiamo infine cercato di proporre il tema dell'ammodernamento della linea ferroviaria Aosta-Torino, della problematica della lunetta di Chivasso, dell'elettrificazione, chiedendo finanziamenti specifici. nel maxiemendamento nulla di tutto ciò è stato recepito, anzi la cosa più spiacevole è che nulla è poi neanche stato discusso. E così, per le politiche della montagna non c'è un posto particolare nei pensieri del Governo. Insisto sulle politiche dei territori montani perché se noi che abitiamo le Regioni alpine non abbiamo strumenti particolari dal punto di vista normativo ed economico, non possiamo pensare di mantenere i servizi alla persona, le scuole, gli ospedali, le micro comunità per anziani e i poliambulatori, nelle nostre bellissime vallate, spesso difficili da vivere, che meritano una sforzo particolare dal punto di vista amministrativo e politico per poter È proprio in quest'ottica che vorrei anche sottolineare come nella manovra vi sia anche l'accordo economico finanziario che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha siglato con il Governo un mese fa circa. Si tratta di un passaggio significativo che si somma agli accordi siglati nelle passate legislature e con le finanziarie scorse, che contribuisce a dare più tranquillità agli enti locali e alla Regione autonoma nel costruire il loro bilancio. In questo accordo la parte sicuramente più importante è la chiusura dei contenziosi in essere, anche se spesso le cifre contenute e il ritorno economico per la Valle d'Aosta appaiono al ribasso e sotto le aspettative. Ciò per far capire quanto sia difficile rapportarsi su questi temi con gli organi del Governo. In conclusione, per ribadire a mia volta e, purtroppo, l'esclusione di fatto del Senato e del Parlamento nel percorso di approvazione di questo disegno di legge di bilancio e la mortificazione delle sue prerogative costituzionali non posso che esprimere un sentimento di preoccupazione generale verso la manovra finanziaria, che contiene tanti interrogativi sospesi, ma soprattutto una forte perplessità sui metodi che il Governo ha voluto seguire in questa delicata e importante fase della vita del nostro Paese.

spazzato i corrotti, festeggiato sui balconi, prolungato i processi a vita, simulato aggressioni subite, fatto scempio della grammatica, sbeffeggiato il sapere, condonato se stessi e gli amici, annunciato bibliche chiusure del commercio, immaginato bambini festosi giocare nelle corsie di emergenza dei viadotti, promesso i soldi i soldi di chi paga le tasse e di chi ha una pensione da 1.100 euro senza implementazione, elevato lo *spread*, abbattuto la borsa, fatto la guerra all'Europa, bruciato 300 miliardi di ricchezza, tassato imprese e automobili, di aver sbagliato, hanno ritrattato tutto, anche male. La sanità è la grande assente e quel poco che c'è è fatto male e con poche risorse neppure certe. Sembra il gioco delle tre carte su quanto c'è per la sanità. riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Sono stanziati 150 milioni per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche. Certamente sono Certamente sono da implementare, ma forse prima serviva pensare di formare il personale che le dovrebbe utilizzare, pensare che tutti i centri potessero essere dotati di banda larga e alla *cyber security*, problema da non sottovalutare. Soprattutto

Magari il Ministro non sa che dovrebbe ricevere un rapporto ogni anno per andare a fondo sui motivi per cui esistono tempi di attesa biblici per fare una TAC o una risonanza magnetica. Per il rinnovo contrattuale e lo sblocco del *turnover*

Il personale sanitario rimane tagliato fuori dai fondi stanziati per i rinnovi contrattuali e sappiamo quanto questo sia necessario, soprattutto per i professionisti delle cure primarie, formati nella gestione del cronico, della complessità, attenti alla salute e alla comunità. Senza un rinnovamento e un miglioramento della formazione dei medici di famiglia non è possibile mettere in atto quanto stabilito anche nel decreto semplificazione.

4 miliardi in dodici anni, dal 2021 al 2032. Ma le formiche negli ospedali ci sono adesso, non aspettano il 2021. Non parliamo dei soliti assenti. Noi abbiamo i nuovi LEA e i nomenclatori tariffari. I nomenclatori non corrispondono a una rubrica con i numeri di telefono delle persone, ma a dispositivi medici impiantati sulle persone, alle protesi che le persone si devono comprare da soli perché il nomenclatore è obsoleto, con dispositivi vecchi, malfatti e pericolosi, che però vengono comunque impiantati, per questioni di risparmio, sui pazienti.

lunga migliore, perché non ci sarebbero le complicanze a cui le malattie croniche oncologiche vanno incontro. Ci volete dire chiaramente quanti sono questi soldi e come verranno utilizzati?

peccato che vengano dati per implementare l'insegnamento della lingua dei segni. Mi sembra di tornare alla scorsa legislatura, quando il Governo Renzi stanziò un milioni di euro,

leggendo il comma 64, in cui si istituisce un fondo pluriennale, con tante belle centinaia di milioni stanziati, per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali. Questo comma rimanda

per le pensioni che oltrepassano il triplo del minimo lordo - si tratta di 1.500 euro lordi mensili - c'è un blocco parziale o anche totale delle rivalutazioni.

ulivi monumentali, esclusi quelli che si trovano nella zona di quarantena, soggetti a radicazione. Praticamente, tutti gli ulivi monumentali centenari sono condannati e non esiste più la tutela che c'era prima, perché fuori dal catasto sono morti, non esistono più.

che si tratta del fulcro della democrazia, perché per gli anglosassoni, - coloro che hanno inventato il parlamentarismo, - non c'è la possibilità di

non interessano i cittadini, soprattutto in questo momento. Tuttavia, si tratta di uno sbrego pesante per la teoria della rappresentanza e la democrazia. Quali sono i rappresentanti con cui avete discusso questa manovra? L'avete fatto con i rappresentanti del popolo in Assemblea? L'avete fatto con i componenti della Commissione bilancio? Forse lo avete fatto all'interno del vostro Governo; nemmeno con i membri della stessa della stessa maggioranza e nemmeno con tutti i membri del vostro Governo. Per un fatto paradossale, forse le persone con le quali avete più discusso questa manovra e con le quali più vi siete confrontati sono quei vertici europei contro i quali avreste dovuto dimostrare la vostra forza. Vi chiedo: ma perché una parte dei cittadini italiani si dovrebbe sentire rappresentata, tra qualche tempo, quando gli effetti di questa manovra si chiariranno? Perché, ad esempio, si dovrebbero sentire rappresentati i cittadini dell'Aquila, ai quali avete negato alcuni emendamenti che non comportavano spesa e altri che avevano copertura? Quando ne ho chiesto conto al commissario, mi è stato risposto che si era trattato di un errore della Ragioneria: i fondi c'erano e ci saranno. Perché quell'errore non è venuto fuori? Perché non vi è stata una sede di confronto. Il vostro confronto si è consumato interamente rispetto alla proposta ideologica che racchiudeva la vostra manovra, quella per la quale non molto tempo fa

del ministro Tria, probabilmente non vi sareste trovati in questo imbarazzo. Cari amici, se da tutto questo c'è da trarre una lezione, c'è da trarre una lezione, è che la sovranità non è un articolo di fede; non è neanche una pretesa ideologica. Rileggete Machiavelli: tutto sommato il vostro Presidente del Consiglio si è comportato pragmaticamente, come i suoi amici i suoi amici contadini della provincia di Foggia, con quella cultura saldamente pragmatica, e probabilmente alla fine ha fatto anche bene.

come l'America di Trump e neanche come altre Nazioni. L'Italia, infatti, è strutturalmente più debole; non è vostra responsabilità e non è responsabilità di questo Governo: la vostra responsabilità è quella di non averlo voluto vedere e, per un tratto ideologico, di aver reso l'Italia ancora più debole. Oggi, infatti, sulla nostra testa

risorse produttive che questa manovra mette in movimento. Peccato che si sia riferito a un solo piatto della bilancia; lui conosce perfettamente l'altro piatto, quello in quello in cui c'è il reddito di cittadinanza, quello in cui ci sono norme sulle pensioni che possono pure rispondere a regole di equità, ma che non sono realizzabili nella situazione di debolezza del nostro Paese. E lui sa perfettamente che quella spesa improduttiva non consentirà la crescita necessaria affinché il nostro Paese non vada in recessione, e sa perfettamente che quelle clausole sono destinate a diventare realtà. Il Il vostro peccato è quello di aver reso l'Italia più debole e forse anche più divisa, perché questa manovra divide ancora di più il Nord dal Sud divide ancora di più le zone interne, soprattutto quelle dell'Appennino meridionale, dalle zone costiere. Voi avete proposto il Governo del cambiamento. Con questa manovra probabilmente sarete i primi ad avere consapevolezza che tra qualche mese sarà necessario cambiare Governo. Noi speriamo che ciò possa avvenire attraverso le regole della democrazia rappresentativa o, magari, anche con un'elezione anticipata, e non attraverso un nuovo sbrego di sovranità, perché qualche straniero viene chiamato qui a riparare i danni che avete fatto per una proposta unicamente ideologica, che non ha nessun contatto con la realtà. Auguri!

il Governo stava consumando uno scandalo parlamentare di dimensioni enormi, non pensavo d'intervenire in questo dibattito. Ho cambiato opinione per quello che ho sentito nella discussione generale e per quello che ho visto nelle ultime ore di questa vicenda. vicenda. Credo che tutti qui, in quest'Aula, abbiano avvertito un sottofondo di spavento un senso di paura per il futuro, una consapevolezza che i nostri destini sono nelle mani di chi considera le regole dello Stato e dell'Europa due fastidiosi ostacoli da abbattere. Questa è la grande questione politica che sta distruggendo il futuro del nostro Paese. L'Italia è governata da forze che non credono nello Stato e non credono nell'Europa. E se, alla fine, Di Maio e Salvini hanno ceduto, certo non lo hanno fatto per spirito europeista, ma per la paura delle conseguenze cui la loro irresponsabilità stava, e sta tutt'ora, esponendo l'Italia. Anche negli interventi dei senatori di maggioranza, depurati dai toni laudatori cui sono obbligati, ho percepito inquietudine e grande incertezza. Persino i toni Persino i toni forti dei senatori Bagnai e Bottici, persino le grida scomposte dei senatori Romeo e Patuanelli nascondevano il disagio di chi è chiamato a difendere una causa che sa essere indifendibile. Ma io avverto nell'aria un elemento politico nuovo, signor Presidente, perché anche molti senatori della maggioranza stanno accorgendosi del *cul de sac* in cui il Governo ha ficcato l'Italia. Anche loro sanno che, nei prossimi mesi, poi per tutto il 2019 e dopo per gli interi anni 2020 e 2021, per l'Italia ogni giorno sarà durissimo, sempre con la spada di Damocle europea sulla testa, sempre alle prese con i controlli e le gravissime condizioni finanziarie cui siamo stati sottoposti in cambio delle mancate sanzioni. Una pace di Pirro che gli italiani pagheranno molto cara. L'Italia ha mostrato arroganza con l'Europa, ha ingiuriato la Commissione, ha predicato un sovranismo eunuco e, come conseguenza, è stata messa in libertà vigilata, non solo dalla Commissione, ma anche da tutte, proprio tutte, le Nazioni dell'Unione europea, compreso Orban, compresa Visegrad, compresa la Lega Anseatica. Quest'anno, né le Commissioni, né l'Assemblea del Senato hanno potuto, non dico votare o esaminare, ma neanche leggere il disegno di legge di bilancio sto intervenendo senza conoscerne nel dettaglio il testo. È per questo che non parlo del merito delle misure, ma solo della dimensione politica del tradimento della democrazia che è in atto.

un testo che è arrivato al Senato due ore fa per essere votato con la fiducia tra poco più di un'ora. Mi rivolgo ai senatori del MoVimento 5 Stelle e della Lega che erano in Senato nella scorsa legislatura: sono certo che si ricordano le urla, gli insulti, il clima surriscaldato, i cartelli, le invasioni dell'emiciclo e persino l'occupazione dei banchi del Governo, con cui tante volte loro stessi protestavano contro una maggioranza che negli scorsi cinque anni mai si era permessa di mortificare e offendere il Parlamento. ieri all'opposizione, oggi in maggioranza, ricordano tutto questo. Lo ricordano certamente e, conoscendo molti di loro, sono certo che sentono il peso non solo delle contraddizioni a cui sono costretti, ma anche della distanza siderale che separa le loro promesse elettorali dalle politiche che Salvini e Di Maio li costringono a votare. Tra poche ore la legge di bilancio tornerà alla Camera. I deputati della maggioranza saranno costretti ad approvarla con la fiducia, ad approvare un testo totalmente diverso da quello che hanno già votato un mese fa. Dopo poche settimane, due voti di fiducia a uno stesso disegno di legge, ma con due testi diversi. E se ci pensate con serenità, colleghi della maggioranza, è una situazione incredibile; in un Parlamento, come il nostro, dove i Regolamenti non consentono di ripetere il voto nemmeno su un emendamento approvato per errore, può accadere che la realtà superi la fantasia. Oggi accade che un disegno di legge venga completamente riscritto e fatto rivotare con la fiducia dopo pochi giorni. Sono certo che quei deputati che verranno chiamati a dare due voti di fiducia su due testi diversi, si renderanno conto di essere stati usati, di non contare nulla e di obbedire a personaggi senza equilibrio, senza esperienza e senza scrupoli. Ecco, osservando i senatori della maggioranza, interpretando i loro silenzi, la retorica dei loro interventi a sostegno del Governo e il loro visibile disagio, si possono incominciare a vedere tra loro delle crepe politiche, dei segni di inquietudine e la preoccupazione di non potercela fare. Questa disgraziata legge di bilancio verrà approvata. L'Italia eviterà l'esercizio provvisorio, ma il trauma di questi giorni avrà effetti politici rilevanti, signor Ministro, soprattutto nella coesione dei Gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega. Politicamente, quel che è accaduto in questi giorni mette la maggioranza su un piano inclinato, segna l'inizio di un percorso di declino, aprirà nei Gruppi parlamentari di Lega e 5 Stelle accesi dibattiti interni, approfondirà il solco tra i due partiti e costringerà il Governo a rendere sempre più esplicito il vero progetto di fondo che questa maggioranza intende propinare all'Italia. È sulla natura eversiva di questo progetto che con il Partito Democratico non è possibile nessuna trattativa. Ieri sera, al centro del bell'intervento della senatrice Bonino, c'era la denuncia dello scandalo di una maggioranza che non perde occasione per indebolire la nostra democrazia parlamentare. Ho molto apprezzato l'intervento della senatrice Bonino, ma con sincerità debbo dirle che lo strame che Governo e Parlamento stanno facendo della democrazia non mi ha proprio sorpreso: l'ho già detto molte volte e lo voglio ripetere. Nel progetto di democrazia diretta che è al centro del programma di Governo (poco fa c'era qui un Ministro che ha proprio questo incarico), il Parlamento è un intralcio che prima va indebolito e poi va abolito. La senatrice Bernini ha ricordato ricordato che Grillo ha detto: «Apriremo il Parlamento come una scatola di tonno». Io non ci trovo niente da ridere in questa affermazione, perché cos'altro vuol dire, come è stato detto, che quando vi sarà un *referendum* alla settimana il MoVimento 5 Stelle potrà anche sciogliersi perché avrà raggiunto il suo obiettivo? anche questo - che fra dieci anni si potrà abolire lo stesso Parlamento che sarà diventato inutile? Cosa vuol dire il Presidente del Consiglio quando si lagna di non poter controllare il Parlamento? Cosa vogliono dire gli attacchi continui dei due Vice Presidenti del Consiglio alla magistratura, alla Banca d'Italia, ai dirigenti del Ministero dell'economia, alle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, alle associazioni di volontariato, alla libera stampa? Signori senatori, tutto è stato chiaramente detto e a nessuno di noi sarà più permesso di dire: «Io non sapevo, io non avevo capito».

prevede che alla fine possano sopravvivere solo due livelli: il popolo e il capo. Ecco, questo è il regime che vogliono per l'Italia e al quale si può dare un solo nome possibile: peronismo (peronismo in salsa Salvini, naturalmente; peronismo in salsa Di Maio).

Davanti allo scempio dell'onore del Parlamento di cui questo disegno di legge di bilancio è solo l'ultimo atto, le Presidenze delle Assemblee non possono più far finta di niente, devo dire con franchezza al Presidente del Senato che il suo richiamo di ieri sera va apprezzato, ma non basta: la ferita è troppo profonda perché tutto finisca così. Rispetto il Presidente del Senato e so che è stata eletta per tutelare e difendere le prerogative della nostra Assemblea e il prestigio dei senatori, ma so anche che solo il presidente del Senato può intervenire non chiedendo, ma pretendendo con la sua autorevolezza che il Senato non venga offeso, umiliato e mortificato. Noi senatori, che contiamo così poco, non possiamo fare un granché; solo il presidente del Senato può dare battaglia dall'alto della sua carica, a favore non di una parte ma dell'intero Parlamento, ricordando a Governo e maggioranza che le istituzioni possono, anzi debbono essere riformate, ma bisogna farlo a viso aperto e non così, spolpandole surrettiziamente come un carciofo, un giorno sconvolgendo le prassi parlamentari e un'altro stravolgendo l'istituto del *referendum*, oppure trattando la riduzione del numero dei parlamentari non come

Zanda. Tra l'altro, credo che la sua argomentazione fosse comprensibile e completa.

sull'umiliazione del Parlamento abbiamo detto molto in questi giorni e in queste della sua mortificazione, che però vorrei dire qui - e spero che anche il senatore Zanda mi ascolti - purtroppo, è una mortificazione

in campo gli anticorpi per ridare forza alla democrazia parlamentare. La tentazione di mettere in disparte i corpi intermedi, di costruire un rapporto diretto tra il capo e il popolo è stata avvertita ed è stato denunciato da molti di noi negli ultimi tempi.

perché rafforzare gli istituti di partecipazione serve non per sostituire la democrazia parlamentare, ma per rafforzarla. Rafforzare gli istituti di partecipazione significa significa ridare forza e voce alla società e ai corpi intermedi e soprattutto rafforzare il Parlamento: esattamente il contrario di quello che abbiamo visto in questi giorni e in queste ore. Qualcuno ha

quando protestavate per le tante fiducie - protestavo anch'io e continuo a farlo - avevate promesso anche questo ai cittadini, nella battaglia referendaria in difesa della Costituzione,

di Liberi e Uguali siamo rimasti fedeli a quella battaglia costituzionale e ribadiamo qui che la Costituzione si difende sempre, non solo quando si sta all'opposizione o quando si scambia la discussione o una battaglia referendaria ampia e istituzionale solo per una battaglia politica. Dico questo nel momento in cui questo Parlamento e quest'Aula del Senato, che noi abbiamo difeso strenuamente anche nella battaglia referendaria,

perché la battaglia sovranista, fatta guardando solo alla propaganda, invece che alla sostanza, ha prodotto ha prodotto il fatto che invece di costruire alleanze in Europa per mettere in discussione quelle regole del rigore che ci hanno strozzati e che hanno prodotto tanta sofferenza in Italia, voi alzate i toni, provocate, non costruite alleanze, forse perché i vostri alleati erano solo e unicamente quelli che erano più rigoristi degli altri. Non avete costruito una strategia - non c'è il senatore Bagnai questa sera, ma in qualche modo lui l'ha detto ieri nel suo intervento - anche nel momento in cui era possibile costruirle, queste alleanze, perché c'era uno scontro aperto tra i vari Paesi. Voi siete riusciti nel miracolo di farli unire tutti contro il nostro Paese. Tutto questo ha portato a un esito disastroso. Volevate fare una prova di resistenza, ma in realtà il cedimento è stato strutturale. La prova di resistenza ha prodotto un cedimento strutturale e l'elemento simbolico più eloquente è l'ordine di Bruxelles di ritardare l'intervento di Conte in Aula perché ad annunciarlo dovevano essere Dombrovskis e Moscovici. Per questo parlo di umiliazione. L'Italia oggi è più subalterna che mai e, soprattutto, siete riusciti nel miracolo di farci legare le mani più di quanto non fosse a settembre e la Commissione ha fatto in modo che fosse assolutamente chiaro. L'Italia sarà d'ora in poi un sorvegliato speciale, tenuto costantemente sotto tiro dalla Commissione con le verifiche - i due miliardi di caparra, tra l'altro, stanno a significare questo

ci hanno ripetuto che le clausole di salvaguardia imposte dall'Europa non significano niente. È una bugia, come dimostra lo sforzo che si è dovuto fare quest'anno per sterilizzare È questa la voce che pesa più e per questo dicevo che siamo legati per tre anni: perché la vecchia clausola era di 13 miliardi, la nuova clausola per il 2020 è di 23 miliardi e per il 2021 è di 28 miliardi.

il *deficit* a zero, né alla flessibilità, avendo già usato quest'anno quella possibile per il triennio. L'accordo capestro con l'Europa ha salvato la vostra propaganda

accordo ha salvato la vostra propaganda, ma solo in cambio di una ghigliottina pronta ad abbattersi di nuovo sul nostro Paese e sui cittadini.

oltre 30 miliardi in meno nel triennio, è ridicolo ed è un insulto all'intelligenza degli italiani. Poi, magari, il ministro Tria ci spiegherà come si potranno fare questi miracoli. La realtà è che questa manovra darà poco a pochi e costerà molto a molti. a molti. Il maxiemendamento non abbiamo potuto esaminarlo in Commissione, ma abbiamo visto le nuove sorprese: ci troveremo ulteriori tagli agli investimenti, altri cinque miliardi di tagli. Esattamente il contrario di quello che avevamo detto. Avevamo detto che per noi il problema non è lo sforamento ma far ripartire il Paese, investire su su un piano verde per fare medie e piccole opere, per costruire occupazione. C'è il rinvio delle assunzioni nella pubblica amministrazione e il blocco della indicizzazione delle pensioni medio-basse. Voi la questione delle pensioni d'oro o di platino, ma intanto andate a spiegare al pensionato, che avrà 1.050-1.100 euro, che ancora una volta dovrà pagare lui. Lo dico al senatore Lannutti: sempre nello stesso modo si fa cassa in questo Paese. tagli per l'editoria - perché vi dà fastidio - che colpirà soprattutto i piccoli giornali. Nel complesso, il Paese alla fine sarà più povero, sia in termini di soldi che di pluralismo e cultura. La cosa più grave della manovra è quello che non c'è: il *deficit* sforato, ma non per un piano di investimenti pubblici capace di creare lavoro e reddito. Non è così solo per il presente ma anche per il futuro. Le clausole accettate implicano che non sarà possibile farlo neppure nei prossimi anni. Vi siete venduti il futuro in cambio della campagna elettorale per la prossima primavera

guardo anche ai banchi del Governo, dove in questi giorni e in queste settimane raramente ho visto una presenza consistente del Governo. Questa sera, questa notte, vedo il ministro Tria e lo ringrazio, perché ritengo che questo Parlamento, che il Senato della Repubblica necessiti di avere un interlocutore e necessiti di essere ascoltato, perché il popolo italiano, i cittadini devono essere ascoltati. una serata, è una giornata, è un periodo che a noi che siamo qui a rappresentare il popolo italiano dà una certa tristezza. Credo che questa sia la volta nella quale il mio intervento avviene con più difficoltà. Faccio davvero fatica, colleghi, a trovare la forza e l'entusiasmo per rappresentare il pensiero che è in me stesso. Lo faccio per il clima politico che ho vissuto in queste due settimane: sono quindici giorni che io e molti altri miei colleghi della Commissione bilancio siamo rimasti qui, incollati al nostro territorio, alle nostre Commissioni e alle nostre sedie, per cercare di apportare un contributo al nostro Paese, però la disillusione è stata totale. Il nostro impegno, la nostra volontà, la nostra caparbietà in certi momenti, non sono serviti a nulla. Le istituzioni che rappresentiamo e loro sì che sono importanti, non noi - purtroppo sono state delegittimate dal comportamento politico di questo Governo e di questa maggioranza.

è qui e che avrebbe dovuto essere, per quanto di nostra competenza, un parere non ostativo oppure ostativo. Ebbene, io mi chiedo come abbiano fatto i colleghi ad avere la capacità di esprimere un parere in dieci minuti su circa 500 pagine di maxiemendamento. Noi di Fratelli d'Italia, per rispetto delle istituzioni, quelle istituzioni che sempre e comunque vogliamo onorare, proprio perché rappresentano il popolo italiano, siamo rimasti seriamente e responsabilmente in sede di Commissione, ma non abbiamo potuto e voluto votare, perché non avevamo gli elementi per esprimere alcun parere, visto che in dieci minuti non era possibile analizzare 500 pagine, tabelle, commi su commi. commi. Questo è il clima nel quale noi oggi siamo arrivati a questa serata. Questo è il clima che mi porta a concludere gli interventi dei miei colleghi di Fratelli d'Italia e che poi porteranno il mio capogruppo, senatore Ciriani, ad annunciare il voto sulla fiducia. La responsabilità, però, ci dovrebbe portare tutti, maggioranza e opposizione, a un comportamento diverso. Non ho apprezzato neppure - e lo dico con quella sincerità che mi appartiene - un certo atteggiamento che il Partito Democratico ha avuto all'inizio di questa seduta. Dobbiamo rispettare le istituzioni; non è urlando o buttando carte per aria che si fa politica. Quindi, come la maggioranza non ha, per me, rispettato il Parlamento, nel momento in cui non ha permesso al Parlamento e alla Commissione di lavorare, ritengo che anche il Partito Democratico non sia stato coerente con quella serietà che il popolo italiano pretende da chi siede su questi scranni. scranni. Credo che ciascuno di noi, al di là dei partiti, debba prima di tutto essere qui non per fare del cinema o del teatro, ma per rispettare se stesso, i propri avversari politici e le istituzioni. Abbiamo il modo di farlo e di dirlo, possiamo dire le cose con forza e e anche con una certa cattiveria, se vogliamo, ma dobbiamo farlo sempre in modo rigoroso e coerente, senza fare sceneggiate, perché il popolo ci guarda, signori. Cari colleghi, il popolo ci sta guardando e, come guarda la maggioranza, guarda anche la serietà con la quale l'opposizione porta avanti le proprie idee. Peraltro, mi sembra anche di ricordare che negli ultimi anni si sia andati avanti spesso a colpi di fiducia, magari non arrivando fino al punto di non far lavorare le Commissioni, ma il malcostume è iniziato da diverso tempo

per il rispetto - lo dico e lo ribadisco - di chi ci ha votato, ma anche di chi non ci ha votato, ma ci vuole interpreti della volontà e della idealità di un Paese intero.

La fiducia su provvedimenti che secondo la nostra opinione non sono stati in linea con quello che serve al popolo italiano.

un provvedimento che rischia, grazie a una demagogia che non ci appartiene, di lasciare sulla graticola per anni dei cittadini magari onesti, ma che si trovano a doversi confrontare con la giustizia. giustizia. Penso alle prerogative costituzionali disegnate dai nostri Padri costituenti, che vengono trascinati per la giacca, perché qui tutti si fanno difensori della Costituzione salvo poi averla tagliata, rigirata e presa a proprio modo, per cui la Costituzione va bene da una parte, però non va bene quando difendeva le prerogative dei parlamentari nei confronti della giustizia, né quando ha portato alla difesa dei vitalizi; cioè sostanzialmente la Costituzione va bene quando va bene per noi e non quando doveva andare bene all'intero arco costituzionale.

di voi nei prossimi anni debba patire le conseguenze di questo giustizialismo demagogico che ha portato il Governo ad approvare quel provvedimento. La fiducia su questi argomenti sicuramente a noi non appartiene,

tramite un parere (che speriamo non venga recepito), voi avete cercato di estendere al diritto fallimentare delle norme che vogliono assolutamente negare la meritocrazia: volete aprire ai consulenti del lavoro l'attribuzione delle

andate a dire ad una cassa privata che si possono condonare i versamenti non dovuti. Le casse professionali, cari colleghi, sono private e come tali vanno rispettate, mentre questa maggioranza che oggi ci chiede la fiducia non rispetta neppure le casse professionali, oltre a non rispettare il merito, come ho detto prima. Fate dei tagli per 38 miliardi nel percorso triennale del disegno di legge di bilancio in esame che investono la produzione di questo Paese.

e se leggete e analizzate le cronache economiche, sapete quanto l'avvicinamento delle aree urbane e suburbane possa aiutare l'economia. Ebbene voi siete contro l'alta velocità,

in vista del 2020, ad una manovra finanziaria già scritta. Avremo le mani legate grazie alla Legge di bilancio che voi oggi, in questa serata, vi attendete ad approvare. Fratelli d'Italia certamente non potrà dare il proprio voto.

in una condizione che ha pochi precedenti, una condizione di strappo istituzionale e di aperta violazione delle regole, come purtroppo abbiamo visto nella seduta di oggi della Commissione bilancio. Una settimana in Commissione a fare finta di discutere della legge e degli emendamenti, senza votarne nemmeno uno. Un maxiemendamento che ha completamente riscritto la manovra che era stata approvata dalla Camera, presentato in enorme ritardo, con errori, fino al pasticcio dell'emendamento sul noleggio con conducente, prima inserito e poi tolto, appellandosi ad un inesistente problema di copertura, per fare poi un decreto, a quanto pare, in una seduta notturna del Consiglio dei ministri. ministri. Personalmente trovo spiacevole che questo importante dibattito, la discussione generale sul più importante provvedimento che assume il Parlamento, non veda l'intervento dei senatori della maggioranza, tra i quali si annoverano molte persone di valore. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ci avrebbe fatto piacere conoscere il loro pensiero, ma evidentemente c'è un ordine di scuderia. Non possono parlare e non possono dire quello che pensano. Non fatevi trattare come delle marionette. Questo è il luogo della democrazia e del confronto delle idee tra maggioranza e opposizione e anche voi avete il diritto e il dovere di dire la vostra. Stiamo discutendo al buio la legge di bilancio, al termine di un percorso gestito disastrosamente. Presidente, se non ci fossero di mezzo i soldi degli italiani, che sono una cosa seria, questo percorso potremmo definirlo una farsa in tre atti. in tre atti. L'avvio del primo atto l'abbiamo tutti bene in mente: la notte del 27 settembre, il balcone di Palazzo Chigi, il vice *premier* Di Maio accompagnato dai suoi Ministri e dalla *claque* di parlamentari e portaborse, che festeggiavano la manovra del popolo,

l'enorme debito pubblico, l'assenza di misure per la crescita, una manovra totalmente sbilanciata sulle spese correnti. Voi, invece, per due mesi avete alimentato nel Paese una grande illusione: illusione: che fosse possibile accontentare tutti, che fosse possibile rispettare un contratto di governo irrealizzabile, l'illusione di finanziare a debito la manovra e di prescindere dall'Europa,

e finalizzato a fare di quello scontro un pezzo della campagna elettorale per le elezioni europee del 2019. Così facendo, signor Presidente, il Governo e la maggioranza hanno lanciato l'Italia a tutta velocità contro un muro, mandando lo *spread* alle stelle, avviando la crescita dei tassi d'interesse per le famiglie e per le imprese, provocando un crollo ininterrotto della fiducia dei consumatori e delle imprese, una fuga di capitali con pochi precedenti e, purtroppo, lo scivolamento del Paese verso la recensione dopo quattordici trimestri di crescita consecutiva. Guardate, prima o poi bisognerà fare i conti su quanto siano costati agli italiani questa follia e questi due mesi di gestione insensata della legge di bilancio. Sono costi che possiamo valutare in miliardi di euro miliardi di euro bruciati in interessi sul debito pubblico e in miliardi di euro di ricchezza dei risparmiatori andati in fumo. Il secondo atto inizia tra il 21 e il 22 novembre. Ministro Tria, il 21 novembre la Commissione europea respinge la seconda versione del documento programmatico di bilancio e avvia i primi passi della procedura di infrazione. Il 22 novembre suona il vero campanello d'allarme: l'asta dei BTP Italia va semideserta, il *flop* peggiore dal 2012, l'allarme vero per un Paese che l'anno prossimo dovrà collocare 400 miliardi di debito pubblico con il rischio che nessuno si compri il debito pubblico italiano, a partire dai risparmiatori italiani. In quei due giorni avete scoperto che il problema più grosso dell'Italia non era nelle stanze di Bruxelles, ma nel nostro Paese, in un muro verso cui avevate lanciato l'Italia e che era molto più vicino di quanto voi stessi vi poteste rendere conto. In quel momento avete innestato la retromarcia e ripreso il negoziato con l'Unione europea, ma l'avete ripreso nelle condizioni peggiori, con un Paese isolato come mai era accaduto in passato. Era isolato rispetto ai grandi *partner* europei, isolato anche nei confronti di quei Governi sovranisti, che teoricamente dovrebbero essere amici di Matteo Salvini e del MoVimento 5 Stelle e che, invece, sono stati i più duri a pretendere il rientro dell'Italia nei parametri europei. I vostri amici e i vostri alleati sono stati i primi a mettervi con le spalle contro un muro e a costringervi a innestare la retromarcia. Vengo, infine, al terzo atto di questa farsa. Il 19 dicembre, due giorni fa, l'accordo con l'Unione europea. Il vice *premier* Salvini - che vedo fare capolino in quest'Aula - aveva con il suo solito tono sprezzante parlato di una letterina di Babbo Natale. la letterina c'è stata, ma è stata quella che il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'economia Tria hanno mandato a Jean Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis dicendo che l'Italia era pronta a tornare indietro sui suoi passi, che la manovra del popolo era uno scherzo e che si andava invece a riequilibrare per rispettare le regole europee. Tutto ciò avveniva nella mortificazione del Parlamento italiano, costretto a fare da spettatore a questa farsa e privato di informazioni essenziali che erano state date alla Commissione europea, ma non al Senato della Repubblica, con tanti saluti alle parole d'ordine sovraniste, alla Repubblica italiana e a una manovra del popolo che dal 19 dicembre non esiste più. Signor Presidente, noi siamo felici che l'Italia abbia evitato la procedura di infrazione. Sia chiaro: noi facciamo sempre il tifo per il nostro Paese. La procedura di infrazione sarebbe stato il colpo di grazia per un Paese avvitato nell'instabilità finanziaria. Gli italiani, però, devono sapere il prezzo altissimo di questi due mesi di follia di follia che saranno costretti a pagare per l'insipienza, il dilettantismo e l'avventurismo con cui è stato gestito il percorso della legge di bilancio. È un prezzo che sta scritto nelle tabelle che vi siete rifiutati di dare alla Commissione bilancio e che finalmente abbiamo potuto leggere. È il prezzo di una manovra che non è più espansiva: è neutra nel 2019 e recessiva negli anni successivi.

le fette di salame sugli occhi e non potrete andare avanti a lungo a raccontare che, con un terzo di soldi in meno, interesserete la stessa platea e con la stessa tempistica a provvedimenti come il reddito di cittadinanza e quota 100. Le nozze non si fanno con i fichi secchi. Signor Presidente, le risorse per la crescita erano già molto limitate nella versione iniziale e il maxiemendamento che ha presentato il Governo riduce le risorse per gli investimenti. Altro che crescita! Questa è diventata una manovra tutta sulla parte corrente ed è una manovra che fa cassa sulle pensioni di 3 milioni di italiani, blocca le assunzioni nella pubblica amministrazione

Sapete quali saranno le conseguenze di questa spada di Damocle? Chi avrà la sfortuna di impostare la manovra per il 2020 potrà fare solo due cose: aumentare le tasse, perché nessuno è in condizione di smontare questa clausola di salvaguardia, e dire agli italiani che abbiamo scherzato e che quota 100 e reddito di cittadinanza sono le promesse di una stagione, buone per le elezioni europee, ma che non ci saranno i soldi

perché l'IVA al 26,5 per cento è un cappio e una spada di Damocle. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Con questa manovra tirate a campare per i prossimi mesi, ma avete compromesso il futuro di questo Paese. Noi non lo accetteremo e voteremo contro, ma saranno gli italiani a non perdonarvelo.

Presidente, vorrei chiarire che anche per il Gruppo Lega è un rammarico che non si sia potuti arrivare in Aula con i relatori e, nonostante questo, penso si possa affermare che il lavoro in Commissione, al di là degli avvenimenti delle ultime ore, non sia stato inutile. Il lavoro è stato utile, sia nell'Aula della Commissione bilancio, sia negli incontri informali e se oggi abbiamo un maxiemendamento, lo abbiamo anche perché i componenti della Commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione, hanno lavorato insieme per migliorare questa manovra. È stata fatta una scelta obbligata, a fronte di una trattativa con la Commissione europea che è durata, ahimè, fino al 19 dicembre. È stata fatta una scelta necessaria per evitare l'esercizio provvisorio ed è stato un tempo utile, perché ha permesso al nostro Paese di evitare la procedura di infrazione. Quindi, dispiace per quanto accaduto, ma abbiamo la certezza di aver fatto tutto il possibile perché il dibattito parlamentare non fosse inutile e avesse una sua utilità. Parliamo dei contenuti della manovra. Innanzitutto per noi era fondamentale riformare la legge Fornero. Era un patto che avevamo preso con i cittadini e che dovevamo onorare. Con questa manovra si fa giustizia per centinaia di migliaia di cittadini che hanno subito una riforma ingiusta e inaccettabile.

Forse sfugge a qualcuno il significato della parola esodati, ma ricordiamo bene che quella legge ha causato anche questo dramma.

Parliamo di una manovra che prevede uno stanziamento di un miliardo di euro per la famiglia, aumenti significativi per il sociale, maggiori stanziamenti per la sanità e l'edilizia sanitaria, la redistribuzione del reddito per le famiglie che più risentono della crisi economica e lo sblocco delle risorse per gli enti locali (dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, al fondo di 400 milioni per i Comuni e 250 milioni per le Province che devono fare manutenzione di scuole superiori e strade).

In poche parole, questa è una manovra che mette al centro equità, giustizia sociale e investimenti per lo sviluppo. C'è poi il capitolo riguardante la trattativa con l'Europa. Qualcuno ha affermato ripetutamente che noi ci siamo arresi, ma ricordiamo da dove arriviamo. Noi veniamo da sei anni di manovre che sono state letteralmente dettate e imposte da Bruxelles. Noi abbiamo invece avviato una trattativa ferma e responsabile. Come tutti ricorderete, nel 2011 un Governo è caduto perché qualcuno voleva imporre la manovra al nostro Paese (gli amici di Forza Italia dovrebbero ricordarselo prima di tutti).

Dopo aver votato quella manovra e la legge Fornero, è ridicolo fare la morale a questa maggioranza e a questo Governo. Governi del PD hanno fatto ancora peggio: avete svenduto il Paese in cambio dell'autorizzazione a spendere in *deficit*; avete autorizzato l'arrivo di centinaia di migliaia di presunti profughi in cambio di flessibilità sui conti pubblici. Questa è la verità.

Sappiamo che molto di più si doveva fare e molto c'è ancora da fare per rimediare a una situazione che è ancora drammatica per la nostra economia e per il Paese. non abbiamo risolto tutti i problemi del nostro Paese - non abbiamo questa presunzione - ma sicuramente siamo orgogliosi di molti dei provvedimenti in essa contenuti.

o poi dovremo porre rimedio. Dispiace poi non essere riusciti a rivedere la norma sulla fatturazione elettronica, che - ricordo - è stata voluta dal precedente Governo, con una copertura di due miliardi

e M5S)*. Siamo tutti consapevoli che per governare serve grande umiltà e grande equilibrio, ma anche grande determinazione e questo Governo sta dimostrando di avere queste qualità. Accettiamo certamente le critiche dei cittadini rispetto a questa manovra; non potremmo fare altrimenti, è normale che accada così. Ma una cosa è certa: non accettiamo lezioni da chi ha sostenuto i Governi degli ultimi sei anni.

da chi ha approvato l'infame legge Fornero, da chi ha svenduto gli interessi del Paese, da chi ha trasformato l'Italia nel campo profughi d'Europa. Non accettiamo lezioni da chi ha arricchito il *business* delle cooperative dell'accoglienza. Non accettiamo lezioni da chi non ha saputo tutelare i risparmiatori truffati dalle banche. Non accettiamo lezioni, in definitiva, da chi ha fallito. *(Applausi dai Gruppi per la crescita del PIL, per il tasso di disoccupazione, per i milioni di famiglie sotto la soglia di povertà. Questo Governo rappresenta una speranza per la maggioranza degli italiani e non intendiamo e non vogliamo deluderli. Vogliamo dimostrare che si può essere orgogliosamente europei, senza essere schiavi di un sistema perverso che schiaccia senza scrupoli i più deboli. Noi non vogliamo un'Europa che, per tutelare gli interessi dei pochi, cancelli i diritti dei molti. Questo è il vostro modello di Europa, non il nostro. Il Governo ha piena legittimità per continuare: ha la fiducia in Parlamento e ha la fiducia nel Paese. Mi rivolgo al Governo: avete dimostrato equilibrio e determinazione, coraggio e senso di responsabilità. Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione si assumerà la responsabilità di sostenere questa manovra e l'azione del Governo del cambiamento. *(Applausi dai che questa non è una manovra perfetta, ma anche la forza e la determinazione di chi ha la fiducia della maggioranza dei cittadini italiani. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Finché sarà così, non saranno certamente le vostre urla in Parlamento a poterci fermare.

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, avrei voluto iniziare il mio intervento sottolineando come, nonostante l'andamento a dir poco discutibile dei lavori d'esame di questo disegno di legge di bilancio, dal confronto parlamentare potesse uscire comunque qualcosa di buono e utile per i cittadini. Invece - ahimè - così non è stato. Vorrei soffermarmi, prima di tutto, su un aspetto del maxiemendamento. Come Come senatore, come Presidente della Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, ma soprattutto come donna e come mamma, è un aspetto che ritengo della massima importanza. Mi riferisco al tema degli orfani per crimini domestici: oggi, nel testo che ci apprestiamo a votare, restano soltanto 5 milioni di euro, a fronte dei 12 milioni richiesti ma soprattutto necessari. Per finanziare, invece, il reddito di cittadinanza, nell'estremo tentativo di riconquistare la fiducia e la fedeltà del vostro elettorato, avete trovato addirittura (ma forse solo sulla carta) 7 miliardi di euro per il solo 2019. Per gli orfani del femminicidio è iniziata in anticipo la stagione dei saldi, ma sul dolore di chi resta non si può e non si deve fare nessuno sconto. Ma veniamo alla vostra sconfitta. Davanti al Paese, nonostante l'ora tarda, avete sollevato volontariamente - o forse inconsapevolmente - un polverone di annunci contrastanti tra loro, per non far capire nulla agli italiani e al Parlamento. Mi chiedo

ma non potete togliere a questo Parlamento il diritto di sapere come il Governo intende spendere i soldi degli italiani. *(Applausi del Parlamento di effettuare questo controllo, viene meno proprio l'idea di rappresentanza parlamentare, viene meno la sovranità del popolo che il Parlamento rappresenta. È alquanto bizzarro che un Governo che si professa sovranista e populista sia poi, di fatto, contro la massima espressione della sovranità popolare. Doveva essere la manovra del cambiamento, ma è stato il cambiamento della manovra! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ci avete concesso soltanto qualche misera ora per decidere le sorti degli italiani. Quindi, vi chiedo se per voi i cittadini italiani valgono soltanto qualche misera ora. Abbiamo fatto insieme a voi, Lega e MoVimento 5 Stelle, nella scorsa legislatura una battaglia comune contro il Partito Democratico che faceva votare provvedimenti a colpi di fiducia notturna. Ma in una cosa siete riusciti: togliere il primato a Renzi! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Voi state emulando il metodo delle *slide*, dei *tweet*, delle promesse cui non seguono i fatti, dell'apparenza e non della sostanza; ma, ancora di più, ci sorprende che state imitando i difetti della peggiore vecchia politica: Ministri e Sottosegretari che si sottraggono al giudizio del Parlamento, misure fantasma, sedute notturne per nascondere i contenuti agli italiani. Ieri gli interventi dei senatori Patuanelli e Romeo mi hanno colpito, perché il loro imbarazzo era talmente palpabile da far risultare il contenuto del loro intervento addirittura imbarazzante. Senatore Romeo (che non vedo),

Quindi, se addirittura il professor Monti, come già annunciato, voterà la fiducia, che ha confermato essere, mai come in questo caso, dettata da Bruxelles, allora sarà più semplice per gli italiani capire in che direzione andrà l'Italia nei prossimi mesi. Di una cosa, però, dobbiamo darvi atto di aver mantenuto la parola: non siete arretrati di millimetri ma di miliardi di euro. Avete fatto un'inversione a U e non siete stati promossi, ma rimandati a gennaio. La procedura di infrazione incombe ancora sulla testa degli italiani. L'Italia rimane un sorvegliato speciale sotto tutela, con tanti saluti al sovranismo. E risulta offensivo nei confronti dei cittadini che il MoVimento 5 Stelle sui *social* e in televisione si vantino di successi inesistenti, che continuino a raccontare menzogne su menzogne, delle quali ormai si è perso il controllo, perché ogni giorno ce ne sono di nuove e diverse che fanno dimenticare quelle del giorno prima. In confronto, la propaganda dell'Istituto Luce era una cosa da dilettanti. E diciamocelo chiaramente: questa manovra è un'enorme *fake news*. È una grave presa in giro per gli italiani che di questa *fake news* si ricorderanno. Mi spiace che non ci sia l'onorevole Di Maio in Aula, perché la sua lista della spesa con le cose fatte la trovo una truffa politica, una grande presa in giro per italiani. Però, visto che tra poco è Natale, forse ha immaginato di scrivere la sua letterina a Babbo Natale con l'elenco dei doni. doni. Avrei voluto, però, dirgli che forse non si è accorto di aver ricevuto in largo anticipo un sacco carico di carbone che scaricherà sulla vita degli italiani. Prima il senatore Renzi è intervenuto citando Abraham Lincoln: «Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre». Ed egli non fa questa citazione a caso, perché lui sa bene cosa significa e ha pagato sulla sua pelle politica le promesse non mantenute. Gli italiani, però, non hanno più gli anelli al naso e, quindi, io vi dico: attenzione, il consenso è come la passione, non dura per sempre, specie se fondato su menzogne. La menzogna più grande e quella più crudele è quella fatta sulle spalle dei nostri pensionati. Avete bloccato la rivalutazione delle pensioni di 1.500 euro. Sono le pensioni dei vostri genitori

In conclusione, non state facendo onore alla Patria, non state rendendo un servigio all'Italia e agli italiani e state invece sacrificando gli italiani

Signor Presidente, colleghe e colleghi, avevo scritto un intervento istituzionale, ma dopo quello che ho sentito e visto in quest'Aula in questi giorni ho stracciato quell'intervento e l'ho riscritto completamente, perché ritengo assolutamente corretto rivolgermi non solo alle colleghe e ai colleghi di quest'Assemblea, ma anche ai cittadini che ci stanno ascoltando da casa, a quelli che a mezzanotte ci sono o ci ascolteranno domani, perché noi non siamo qui per fare lo *show* televisivo nei confronti degli italiani, ma per mandare avanti questo Paese, e poco importa se votiamo a mezzanotte, alle 5 o alle 10 di mattina.

E non avrebbe potuto essere diversamente visto il disastroso quadro economico e sociale che abbiamo ereditato dai precedenti Governi, e quindi abbiamo il dovere di imparare dagli errori del passato. Credetemi che qui abbiamo un ampio bagaglio da consultare per poter migliorare questo Paese. Questa viene chiamata manovra «del» popolo, ma più correttamente la definisco la manovra «per il» popolo, perché è per il popolo che la stiamo facendo. *(Applausi È il voto popolare che stiamo onorando e rispettando e noi siamo sempre qui in Aula, al contrario di quei senatori eletti che invece qui non si fanno mai vedere,

proprio quel rispetto delle istituzioni che una collega ieri ci ha detto che non abbiamo e che invece rivendico con orgoglio, perché se siamo qui in quest'Aula è proprio per il rispetto delle istituzioni e l'amore per il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e* *L-SP-PSd'Az).* Siamo qui per cercare di rimediare agli errori di tutti quelli che hanno governato l'Italia negli ultimi trent'anni e che l'hanno messa in ginocchio. Perdonatemi un altro inciso sulla questione del rispetto: se vogliamo ricevere rispetto, in quest'Aula e fuori di qui, dobbiamo esseri prima di tutto noi a rispettare gli altri, perché il rispetto non parte dalla testa, ma da noi stessi. Pertanto mi auguro che qui in futuro nessuno più si possa permettere di indirizzarsi al Presidente del Consiglio dei ministri,

Come è mancanza di rispetto delle istituzioni dire al Presidente del Senato che oggi siete andati a «consegnare dei fogli» al Governo - quelli della manovra - quando abbiamo visto tutti chiaramente che sono stati lanciati in aria, con un *pièce* teatrale mi auguro non sia andata in onda, e non per la vostra immagine, ma per il basso livello di rispetto delle istituzioni che state dimostrando al Paese.

Dicevo, questa manovra è per il popolo ed è la prima volta che con una manovra si pensa davvero a chi in questo Paese non viene considerato, a chi esce dal mercato del lavoro e non sa come rientrare, a chi vuole cominciare a lavorare nella legalità, ma non ce la fa per i mille lacci e laccioli che imbrigliano i nostri imprenditori e liberi professionisti, a chi vorrebbe andare in pensione dopo una vita di lavoro e non può farcela per colpa di una legge che ha innalzato i limiti di età. Parliamo di fiducia sulla manovra. Partiamo dalla Comunità economica europea, che poi è diventata Comunità europea e infine Unione europea: Comunità, che poi diventa Unione, e il termine «economica» che scompare via via, segno che l'intento era di creare un insieme di Nazioni che partisse dagli aspetti economici per poi arrivare, nel tempo, a essere una unione di Nazioni liberamente aggregatesi. Per unificare le Nazioni si è partiti unificando quell'elemento comune più semplice da gestire, la moneta, che è stata il *driver* che in tutti questi anni ci ha gestiti. L'euro doveva essere il primo passo, il più semplice da gestire e importante per unire questi Paesi; il fattore abilitante per fare tutto il resto e migliorare la vita di tutti. di tutti. «Con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più», ricordate? Ma ci si è praticamente fermati lì, e non lo dico con cattiveria, chiariamoci, ma perché chi ci ha malgovernato in questi anni ha ritenuto che fosse sufficiente gestire l'aspetto economico per poter unire davvero i popoli.

Paesi che sono andati in *default* o quasi, come Grecia e Portogallo, e per quanto riguarda l'Italia 5 milioni di poveri sotto la soglia della povertà assoluta. Mi dispiace che in quest'Aula si citi molto spesso il falso, dicendo, per esempio, che si vanno a ridurre le pensioni da 1.300-1.500 euro.

O, peggio ancora, quando qualcuno che ha guidato questo Paese ha detto che il reddito di cittadinanza costa 63 miliardi di euro: ma dove lo ha letto? E poi subito dopo ha detto: «Avete mentito, avete truffato gli italiani». Qui chi mente agli italiani è chi ha promesso, dopo aver perso il *referendum*, di andarsene a casa e invece è seduto in quest'Aula.

Dopo la terza censura si vince il premio! DELL'OLIO *(M5S)*. Tra l'altro, ha anche detto che il presidente del Consiglio Conte è andato a patteggiare con l'Unione europea; ma se il presidente Conte ha patteggiato - come dice lui - per evitare di far andare in infrazione l'Italia, e quindi per il bene dell'Italia, lui invece ha svenduto l'Italia quando è andato a farsi autorizzare gli 80 euro per una necessità elettorale. Cosa c'entra questo con la fiducia? C'entra, perché la fiducia che i nostri passati Presidenti del Consiglio hanno fatto venir meno da parte dell'Europa nei nostri confronti è fondamentale per la sopravvivenza del nostro Paese nell'Europa stessa. Quindi, ecco che invece la capacità del presidente Conte, e di tutto il Governo, di affrontare una complessa trattativa con l'Europa si è tradotta in un risultato eccellente: quello di riuscire a evitare la procedura di infrazione, senza che il Governo dovesse rinunciare alla filosofia ispiratrice e alle misure di investimento sociale che caratterizzano la legge di bilancio. Questo è un passo - e neanche tanto piccolo - verso la direzione di riguadagnare la fiducia in Europa e di dare a noi italiani un motivo in più per dare fiducia a questo Governo. Dal prossimo anno possiamo mettere in campo il reddito di cittadinanza, il superamento della legge Fornero, l'aumento delle pensioni minime, il riconoscimento dei sacrosanti diritti dei risparmiatori traditi dalle banche,

con questa manovra abbiamo il merito, e siamo orgogliosi di aver dimostrato, anche alla Commissione europea, che mai come oggi è necessario mettere a fuoco che la stabilità finanziaria, quella tanto cara a Bruxelles, non può essere più scissa dalla stabilità sociale. L'Unione europea che verrà, quella che in primavera verrà rinnovata nei suoi organi, che nel tempo ha lasciato indietro troppi cittadini, sarà senza ombra di dubbio un'Unione europea con un ampio punto di vista sul sociale e, finalmente - ce lo auguriamo tutti - diventerà davvero un'Europa unita, non più solo formalmente per via della moneta, ma di fatto perché le politiche sociali - interne e comunitarie - verranno affrontate e gestite dando a ogni Paese il giusto spazio per migliorare economicamente e socialmente. Il MoVimento 5 Stelle e la Lega, quando hanno firmato il contratto di Governo, un altro segno di rispetto delle istituzioni (non certo un patto del Nazareno nascosto o altri inciuci, ma un documento liberamente consultabile da tutti), lo hanno fatto inserendo oltre 30 punti da portare avanti nella legislatura: oltre la metà di questi punti sono stati affrontati in questa manovra ed è solo la prima. È una manovra perfetta? No, certo, sempre e comunque si può migliorare, e avremmo voluto fare sicuramente di più e meglio, ma data la situazione disastrosa in cui abbiamo trovato questo Paese, e la spada di Damocle della procedura

e la regola del debito era solo il capro espiatorio; la seconda è che quando parliamo della sterilizzazione delle clausole dell'IVA, come è stato già detto dalla collega Bottici, occorre ricordare che dal Governo Monti in poi queste clausole sono sempre state previste, con gli impegni di ogni Governo a sterilizzarle per l'esercizio successivo, e proprio il senatore Monti, parlando di polvere sotto il tappeto, anzi di tappeto volante, ne ha assunto la responsabilità dicendo - testualmente - che questa situazione «in parte l'abbiamo costruita noi». Quindi, cara opposizione, se volete prendervela con qualcuno, per una situazione che nel tempo è peggiorata, non gridate «al lupo, al lupo!» ma mettetevi una mano sul cuore e l'altra sulla bocca, e non parlate più di questo argomento.

Il MoVimento 5 Stelle ha fortissimamente voluto sia l'adeguamento dei vitalizi dei parlamentari sia il taglio delle pensioni d'oro. E questo è solo l'inizio, per cui volendo prendere i punti...

e questo è solo il primo passo verso il cambiamento che questo Paese aspettava da molto, troppo tempo.

Signor Presidente, signori membri del Governo, cari colleghi, il MAIE - Movimento Associativo degli Italiani all'Estero è presente in Parlamento dal 2008 la prima volta constatiamo che una maggioranza di Governo realizza quanto è stato promesso in campagna elettorale. Come italiani all'estero, siamo orgogliosi di un Governo che difende gli interessi del nostro Paese, conciliandoli in maniera intelligente con l'Europa. Nel merito delle misure di nostro diretto interesse quali italiani all'estero, intendiamo apprezzare in particolare la decisione di autorizzare l'incremento in 350 unità del personale assegnato alla rete consolare (300 unità di personale di ruolo

da un lato, si conferma un impegno contenuto nel contratto di Governo al punto 10; dall'altro, consentendo di migliorare i tempi dei servizi consolari, è una misura decisiva per combattere efficacemente quella che possiamo definire la "mafia degli appuntamenti". È così e lo ripeto: la mafia degli appuntamenti. Quella rete di intermediari che, benché contrastata dai Consolati, si è sviluppata negli ultimi anni e impone a tanti connazionali il pagamento di cifre assurde per poter accedere a un servizio cui hanno diritto, al rinnovo del passaporto o pratica di cittadinanza. Inoltre, vorremmo sottolineare il fatto che questa legge preserva la stampa italiana all'estero, un servizio che oltre a dare informazione, promuove la nostra lingua, la nostra cultura e il *made in Italy*.

Signor Presidente, in queste settimane abbiamo visto cose che speravamo di non dover vedere. Prima il balcone di Palazzo Chigi, poi il conflitto con le istituzioni europee, lo *spread* che aumentava, la Camera costretta ad approvare una legge di bilancio provvisoria, la promessa che il Senato avrebbe avuto modo e tempo di lavorare sulla manovra. Per giorni siamo rimasti in attesa dell'accordo con l'Europa. Poi è venuto il Presidente del Consiglio in Aula ad annunciare che non ci sarebbe stata la procedura d'infrazione. Noi abbiamo espresso il nostro sollievo e abbiamo detto: «Adesso però fateci lavorare». In Commissione c'erano migliaia di emendamenti e maggioranza e opposizione avevano già fatto una cernita dei più importanti, proprio per dimostrare spirito di collaborazione. Intanto, però, il maxiemendamento non arrivava, ma arrivava invece la peggiore delle decisioni, quella del testo presentato direttamente in Aula. Lo dico a beneficio di chi ci guarda da casa: vuol dire che tutte le proposte, tutto il lavoro preparatorio della Commissione, tutti i confronti, le segnalazioni, le riformulazioni riformulazioni valevano quel che valevano: poco. Come bisogna anche dire che è inutile anche perché con la fiducia non c'è nessuna possibilità di dialettica parlamentare e di modifica del testo, ma solo la possibilità di prendere o lasciare. Sono state messe in fila una serie di forzature senza precedenti; in tanti anni vissuti nelle istituzioni locali non avevo mai visto nulla del genere. Noi ci uniamo alle parole che la presidente Alberti Casellati ha espresso ieri in quest'Aula al grido d'allarme lanciato dal presidente Napolitano. Il Senato non può essere trasformato in una sala d'aspetto. Il Senato non può essere privato delle sue funzioni e delle sue prerogative. Il Senato non può essere umiliato in questo modo.

che per noi la democrazia parlamentare è l'unica garanzia per una minoranza, perché è essa che ti costringe a trovare il compromesso ti costringe a trovare sempre la soluzione nella moderazione e non nelle posizioni estreme. *(Applausi che garantisce anche una minoranza linguistica come la nostra. Quindi mi fa paura se vedo che la democrazia parlamentare viene così umiliata. Noi non avevamo pregiudizi su una manovra espansiva, che, a costo anche di qualche forzatura, puntasse con decisione alla crescita e allo sviluppo. Invece qui, nonostante i tanti annunci, non solo la crescita viene dimenticata, ma la pressione fiscale non diminuisce e rischia di alzarsi sia per le imprese, che per le famiglie. Se l'Italia fosse una famiglia si potrebbe ben dire che le sono state fatte firmare una montagna di cambiali, che andranno onorate nel volgere in pochi mesi. Le clausole di salvaguardia penseranno come macigni sull'attività del Governo: 23 miliardi di euro da trovare entro il 2020 e 29 altrimenti l'IVA schizzerà prima al 25 e poi al 26,5 per cento. Non voglio adesso continuare su questa tematica, perché chiunque, qui e anche fuori, tutti i cittadini sanno cosa voglia dire per i consumi se l'IVA aumenta al 26,5 Sulle misure chiave noi la pensiamo così. Il problema delle pensioni non può essere inquadrato solo dal punto di vista di chi vuole andare in pensione, ma anche da quello di chi pagherà quelle pensioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Difficilmente quota 100 aiuterà il *turnover* nel mondo del lavoro. Lo dicono tutti, lo spiegano le ricerche: l'automatismo tra una persona che lascia il lavoro e una che entra non esiste. Sul reddito di cittadinanza scommettete sul fatto che i centri per l'impiego sapranno dare un lavoro a chi non ce l'ha; ma il lavoro lo creano le imprese e in questa manovra secondo me

assistenzialistica, che favorirà addirittura, se non fate attenzione, il lavoro nero. Lo abbiamo detto con forza in queste settimane: mettete al centro la crescita e lo sviluppo. E invece scopriamo che avete congelato 650 milioni di euro a favore del sistema produttivo con la clausola di salvaguardia in uscita; avete cancellato gli investimenti su ferrovie e cantieri; avete destinato appena un miliardo all'innovazione, quando un Paese come la Francia nel 2016 ne metteva 10; avete cancellato 850 milioni per le politiche comunitarie, con il rischio di rallentare l'esecuzione dei progetti finanziati per il 2019 all'interno della programmazione 2014-2020; avete ridotto le agevolazioni fiscali per gli enti non commerciali, ossia le attività di volontariato, di assistenza sociale e di impegno nel sistema socio-sanitario. Con la *web tax* sono in molti a dire che a pagare non saranno i colossi della rete, come sarebbe giusto, ma soprattutto le piccole e medie aziende italiane che hanno costruito piattaforme di vendita digitale. Ci sono poi i tagli ombra per gli enti locali, a cominciare dal rinvio delle assunzioni per la pubblica amministrazione. Vede, signor Presidente, è difficile essere contenti quando una legge di bilancio, che nelle intenzioni doveva restituire risorse ai cittadini, rischia di fare l'esatto opposto. Noi siamo sollevati - e lo dico con sincerità - per il fatto che sia stata evitata la procedura di infrazione; e lo saremo anche quando saremo certi che si eviterà l'esercizio provvisorio. Ma questo sollievo non può cancellare le fortissime perplessità per una manovra che non ha respiro, che scommette tutto su due misure bandiera e sulla quale probabilmente anche alla Camera verrà posta la questione di fiducia. Questa manovra è una nube nera sull'economia italiana. Per il bene dell'Italia, speriamo che la tempesta non scoppi mai, ma è molto difficile; è molto difficile non sentirsi pessimisti. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Per le Autonomie alla legge di bilancio.

colleghe e colleghi, abbiamo avuto a disposizione il disegno di legge di bilancio alle ore 16 di quest'oggi e fra qualche decina di minuti la voteremo. È un record storico: mai è accaduta una cosa del genere. La Camera ha votato la fiducia su una manovra finta; la Commissione non ha potuto discuterne e affrontarla perché la manovra non si conosceva. Come ha detto il senatore Quagliarello a ragione, forse nell'immediato non interessa molto ai cittadini italiani,

i burocrati della Ragioneria generale dello Stato; ma quand'è che vi assumerete la responsabilità di essere Governo di questo Paese? Quando ve la assumerete questa responsabilità? Non vi sfiora nemmeno il fatto che di fronte ai tempi così stretti avreste dovuto chiedere chiedere a quest'Assemblea di fare uno sforzo e le minoranze vi avrebbero detto di sì. No, schiaffi e schiaffoni, perché tanto questo è l'unico linguaggio: schiaffi e schiaffoni. Ma questo non è il problema. Il racconto che è colpa di questi o di quelli si infrangerà nella verità. Avete affrontato la trattativa con l'Europa; è un fatto assolutamente positivo che non ci sia la procedura d'infrazione, almeno per ora. Quindi, bene presidente Conte, ma

sapevate tutto già da prima, vi bastava ascoltare il ministro Tria, che due mesi fa vi aveva detto come stavano le cose. Tutti i centri internazionali, europei e mondiali ci avevano spiegato che l'economia stava prendendo un'altra strada, così come sapevate che i mercati non si sarebbero impressionati dalle dichiarazioni di Di Maio e di Salvini. I mercati non si impressionano delle delle dichiarazioni di Di Maio e Salvini: i mercati le ascoltano e scelgono di colpire l'Italia ed è quello che è successo. Voi siete partiti per suonarle all'Europa e siete stati suonati dall'Europa. Qualcuno di voi ha detto: «Me ne frego». Sì, ma a sbattere c'è andata l'Italia. Voi ve ne potete fregare, ma i risparmiatori, le imprese, le famiglie italiane purtroppo non se ne possono fregare.

Non avete chiesto, come sarebbe stato utile per il Paese, al Parlamento italiano. Assumiamo una posizione insieme, andiamo in Europa e chiediamo di cambiare le regole che non condividiamo, che non vanno bene, che sono recessive. non avete fatto questo. Voi avete dato schiaffi, schiaffoni e ne avete presi tanti, ma non avete chiesto. Noi vi avremmo dato il nostro sostegno per andare in Europa a chiedere, dopo quanto è accaduto (Genova, le alluvioni, il rapporto

con il voto di questo Parlamento e avrebbe avuto la forza per provare a cambiare qualcosa. No, non avete fatto questo e avete compiuto un grave errore, che il Paese paga e soprattutto pagherà. Potevate chiedere e proporre. Senatore Bagnai, lei dice sempre cose intelligenti e io la ascolto sempre con grande attenzione, ma non non una traccia di un'iniziativa politica del Governo per cercare di costruire un altro rapporto con l'Europa. No, voi avevate bisogno della spesa corrente corrente e di finanziare quota 100 e reddito di cittadinanza. Siete andati dritti per quella strada e qui il paradosso: vi siete isolati prima di tutto dai Governi dai Governi sovranisti che sono stati i più duri a chiedere di punire l'Italia. Sento adesso qualcuno dire che arriveranno le elezioni europee

in due anni. Chi la farà la manovra? Quanto dovranno pagare gli italiani? Questo è il problema, questo è il punto; vi siete messi in un vicolo cieco in nome della demagogia fatta dal popolo a sua insaputa.

soffermarmi ancora su un punto che mi interessa molto. Ciò che sta succedendo frutto dell'inesperienza. Non ho mai detto e non dirò mai che siete degli incapaci. Io i miei avversari politici li rispetto. Io temo qualcosa di più serio. Temo che qui ci sia un'idea di democrazia o di democratura che va nella direzione nella direzione di Orbán, Putin ed Erdoğan. Vi prego di pensarci; la democrazia senza bilanciamenti, l'insofferenza per gli enti enti autonomi, Banca d'Italia, magistratura, qualsiasi ente autonomo, è un problema per l'Italia e per la qualità della sua democrazia. Questa legge non l'hanno fatta i malati. Voi prevedete un aumento di un miliardo, già annunciato dal Governo Gentiloni Silveri, che non è nemmeno sufficiente a coprire il contratto del comparto e i livelli essenziali di assistenza bloccati al MEF. Non è nemmeno sufficiente questo. Non c'è il taglio del superticket, che è un *boomerang* anche economico nei confronti del Servizio sanitario nazionale. I medici fanno sciopero. La povertà

e non troveranno lavoro. Sovrapporre il reddito di cittadinanza con la questione del lavoro è un gravissimo errore. Voi avete fatto una manovra

mettendo prima di tutto davanti gli italiani, le imprese che pagheranno più tasse, il fatto che non c'è un'idea di sviluppo e di crescita, una politica industriale e una visione. Noi Noi daremo un voto contrario a tutela degli interessi dell'Italia e di tutti gli italiani.

probabilmente per la prima volta nella sua storia il Senato si accinge a votare una manovra di bilancio che non ha letto, non ha potuto emendare, non ha potuto studiare e non ha potuto nemmeno tentare di migliorare. La responsabilità di questo *vulnus* istituzionale piuttosto grave ricade sulle spalle del Governo e della maggioranza. Non ci sono scuse accoglibili sotto questo profilo. la verità, purtroppo, è che i dettagli, anche minimi, di questa manovra li conoscono il signor Juncker e il signor Moscovici, ma non li conoscono i senatori della Repubblica italiana. *(Applausi Per cortesia, evitateci le scuse che abbiamo ascoltato in questi giorni in Aula e nei comunicati stampa del Governo e della maggioranza, che vorrebbero farci credere che il ritardo imbarazzante con cui avete consegnato il maxiemendamento è una dimostrazione della vostra autonomia rispetto ai *Diktat*

per decidere come riempirli perché i soldi sono pochi e le promesse tante, probabilmente troppe. Presidente Conte, noi in quest'Aula più volte - e lo ribadiamo ancora in questa occasione - abbiamo detto che avremmo fatto un'opposizione responsabile, leale

la tragedia dell'esercizio provvisorio, sarà grazie al senso di responsabilità dimostrato dalle opposizioni all'interno del Senato della Repubblica e, in particolare, grazie alla responsabilità che noi abbiamo dimostrato

Vi abbiano chiesto - potrei dire che vi abbiamo scongiurato - di non rendere obbligatoria la fatturazione elettronica, che ha l'unico scopo di incassare due miliardi di euro dal portafoglio di commercianti e artigiani, che già adesso fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, ma è stato tutto inutile. Vi abbiamo proposto di ragionare insieme sul quoziente familiare, vi abbiamo ribadito la nostra proposta della *flat tax* incrementale, che non costa nulla e che garantirebbe incassi allo Stato. Vi abbiamo proposto di ragionare intorno alla riduzione del cuneo fiscale,

disatteso. Presidente Conte, colleghi della maggioranza, ribadiamo che tutto il male che pensate della Commissione europea e dei dieci anni di rigore, noi lo pensiamo moltiplicato per due, per tre, per cinque o per dieci volte, perché la politica che ha seguito l'Europa nell'ultimo decennio è stata la politica della sordità rispetto al fatto che il ceto medio si è impoverito. La Commissione europea, composta da euroburocrati, è stata sorda rispetto al dolore dei ceti sociali colpiti dalla globalizzazione.

per un piano straordinario di investimenti, sia pubblici che privati, per la manutenzione del nostro Paese, per investimenti ad alta tecnologia, che sono il futuro dell'Italia, saremmo stati al vostro fianco fino all'ultimo respiro. Il problema è che, dopo mesi di battaglie annunciate, di guerre giornalistiche e poi di ritirate sufficientemente vergognose, tutto questo *caos* che avete creato, al di là degli effetti sullo *spread*, sui risparmi e sulla borsa, serviva ed è servito ad un unico obiettivo politico: garantire al MoVimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza e garantire quindi la possibilità di sventolare una bandiera elettorale, per quanto ormai logora e bucherellata, perché il reddito di cittadinanza non sarà certamente quello promesso in campagna elettorale. Questa è la semplice e triste verità. Tutto l'impegno che avete profuso per una finta guerra con l'Unione europea serviva semplicemente e solo a poter annunciare dal balcone di Palazzo Chigi - beati voi! - la cancellazione e l'abrogazione per legge della povertà e per poter annunciare dagli schermi televisivi la consegna di sei milioni di tessere prepagate per il reddito di cittadinanza, da consegnare ad altrettanti cittadini ed elettori. Vi siete assunti la responsabilità

Presidente, devo ricordare che qualche giorno fa, a un convegno organizzato da una fondazione di destra, il sottosegretario Giorgetti, probabilmente voce dal sen fuggita, ha detto che il reddito di cittadinanza piace all'Italia che non gli piace. Il problema è che voi, alla fine, lo voterete e noi non lo voteremo. Lo voterete nonostante siate assolutamente consapevoli dei danni che provocherà, sia in termini sociali che in termini economici, per i suoi effetti recessivi. Dov'è finita la manovra espansiva, primo ministro Conte e ministro Tria? Facciamo davvero fatica a vederla. Dove sono finiti il taglio delle tasse e la *flat tax*? non raccontateci che la *flat tax* è l'aumento del regime forfettario, che riguarda poche centinaia di migliaia di persone, a fronte di milioni e milioni di partite IVA e di imprenditori che vedranno le tasse

Noi vediamo soltanto un cortocircuito, fatto da più tasse, meno investimenti, un PIL che cresce in maniera striminzita, più debito e, soprattutto, più sfiducia da parte dei consumatori e delle imprese. Il fatto più grave, anche se è il più difficile da spiegare ai cittadini e a chi ci ascolta, è la vostra decisione di sottoscrivere le clausole di salvaguardia, che valgono 50 miliardi miliardi di euro nei prossimi due anni. Rispetto a queste, quelle previste dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri sono acqua fresca. Presidente Conte, credo che lei si renda conto che voi avete deciso di commissariare il nostro Paese. Vi siete autocommissariati, perché chiunque avrà l'avventura di governare l'Italia nel dicembre dell'anno prossimo si troverà a partire da meno 23 miliardi di euro, a cui facilmente dovrà aggiungere il mancato gettito derivante dalle dismissioni dei beni pubblici.

prossimi anni, perché chiunque governerà non potrà avere la minima libertà fiscale, né sociale. Il prossimo bilancio lo scriveranno i funzionari del Ministero, perché, una volta coperte le spese obbligatorie e correnti, non ci saranno più soldi per nulla. La narrazione politica con cui ci avete ossessionato con cui ci avete ossessionato negli ultimi anni - quota 100 e reddito di cittadinanza - non descrive l'Italia vera. Sembra che l'Italia sia divisa tra chi vuole andare in pensione, legittimamente, in anticipo e smettere di lavorare

Gli riconosciamo il fatto che lo ha fatto da solo, perché coloro che hanno dichiarato guerra all'Europa si sono tenuti ben lontani dal campo di battaglia al momento della resa, dell'umiliazione e del compromesso.

collaborativo, ma abbiamo trovato di fronte un muro. La manovra che voi approvate non è quella che avevamo immaginato e sognato e - soprattutto - non è quella per cui abbiamo chiesto il voto ai cittadini.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, autorevoli Ministri e rappresentanti del Governo, cari colleghi, sono state settimane, giorni e ore molto difficili in quest'Assemblea. La ferita è profonda. Noi riteniamo che il Senato della Repubblica e il Parlamento italiano siano stati continuamente offesi dal vostro atteggiamento, dal vostro modo di fare e dal vostro modo di intendere la politica. Signor Presidente del Consiglio, è la prima volta nella storia della Repubblica che viene fatto un disegno di legge di bilancio totalmente e completamente extraparlamentare, che non ha permesso alle Commissioni tutte, in particolare alla Commissione bilancio, come previsto dalla Costituzione, di approfondirlo. Lei, signor Presidente del Consiglio, ci ha messo del suo: suo: è arrivato a dichiarare che era dispiaciuto di non poter controllare il Parlamento; ma lei, che è un autorevole professore, sa che esiste la divisione dei poteri, sa che il Parlamento è autonomo, sa che il Parlamento ha dei diritti. PD* *e FI‑BP)*. Signor Presidente del Consiglio, credo che lei, il suo Governo, i suoi Vice Presidenti, i suoi Ministri questi diritti, in queste settimane, li abbiate più volte calpestati. Credo che si sia usata della violenza, nelle ultime ore anche fisica, ma, nell'arco di questi giorni, sicuramente violenza politica da parte vostra. Avete avuto atteggiamenti molto pesanti; avete volutamente, con intenzione, con metodo, fatto in modo che le nostre Commissioni, il nostro Parlamento, i nostri parlamentari,

sono stati fugati in Assemblea pochi minuti fa. Ringrazio il senatore Tosato e il senatore Dell'Olio, perché il loro intervento ha testimoniato, con chiarezza, con trasparenza, in maniera limpida, che neanche i senatori di maggioranza conoscono la manovra. *(Applausi dai Gruppi PD* *e FI-BP)*. Ne hanno fatto una descrizione irreale; non posso dire falsa, perché non conoscevano la manovra, ma hanno dimostrato quello che è incredibile, incredibile, impossibile in una democrazia parlamentare. Quello che avete fatto è molto, molto grave. Ho apprezzato molto le parole della senatrice Bonino, Bonino, perché ci ha messo in guardia dai vostri comportamenti, dal vostro modo di essere e dal vostro modo di intendere la politica. Badate bene, avete sbagliato anche nel porvi nei confronti della Commissione europea: ci avete ridicolizzato, avete ridicolizzato il Paese. PD)*. Ricordo le parole del vice *premier* Di Maio dal balcone, quando ha abolito la povertà. Molti italiani ancora si interrogano su questo. Ricordo anche le parole del vice *premier* Salvini, quando ha detto che non si sarebbe mai arretrato dal 2,4 per cento di*deficit*. Mi domando: chi rappresentavano nel momento in cui parlavano? Rappresentavano, signor Presidente del Consiglio, il suo Governo?

strafottenti; ricordando D'Annunzio (dimostrando anche che i nostri Vice *Premier* hanno una cultura adeguata al ruolo che ricoprono), hanno detto che loro se ne sarebbero fregati dello *spread*, che lo *spread* non interessava a nessuno. «Io me ne frego», sono state le parole dette testualmente dal presidente Salvini. Perché «Io me ne frego»? Perché i denari,

E poi anche le offese. Mi ricordo anche le offese. Le offese del presidente Salvini al presidente Juncker. Mi dispiace che il presidente Salvini non sia in Aula, ma bisogna stare attenti. Non è corretto e non è giusto, anche da un punto di vista etico, offendere le persone per dicerie, anche perché le dicerie riguardano tutti.

Noi non offendiamo le alte cariche istituzionali, né internazionali, né europee, né italiane. E forse il presidente Salvini da lei, Presidente del Consiglio, dovrebbe essere richiamato ad avere rispetto istituzionale e personale. Ribadisco: tutti hanno qualcosa da nascondere. Ricordiamocelo. Era forse un modo per distogliere l'attenzione dalle tante bugie? Allora, ricordiamo il vice presidente Di Maio, con quell'elenco divertente di *fake news* e di bugie su cose fatte. Io ho una lista diversa delle cose che voi avete fatto, signor Presidente. Voi avete certamente, dopo il decreto dignità,

Voi, signor Presidente del Consiglio, con il decreto sicurezza, voluto dal vice *premier* Salvini, avete sicuramente aumentato il numero delle persone non regolari e sicuramente avete aumentato l'illegalità in questo Paese:

di avere un Paese più insicuro, un Paese che abbia paura, un Paese che richiami e richieda l'ordine. Questo fa parte di un disegno pericoloso che lei, il suo Governo e i suoi Vice Presidenti state portando avanti! E poi c'è questa manovra. Questa manovra disastrosa, pericolosa per il futuro del nostro Paese, sulla quale continuate a raccontare in maniera metodica, continuativa, con grande determinazione, molte bugie. bugie. Ci sono le imprese che faticano e voi che aumentate le tasse. Ci sono le esigenze della macchina pubblica e voi che bloccate il *turnover*. C'è la cultura, la scuola, l'università, la ricerca, che voi penalizzate con grande forza e determinazione. Non sarà un caso. Poi ci sono gli altri provvedimenti, con l'accanimento nei confronti dei pensionati che prendono 1.500 euro lordi, signor Presidente: 1.500 euro lordi! Voi bloccate loro gli aumenti. Voi li volete penalizzare e volete finanziare i vostri assurdi provvedimenti con i soldi dei pensionati. Io credo che questo sia davvero molto grave! Non parliamo dell'IRAP, ma parliamo, per esempio, del volontariato al quale voi avete raddoppiato le imposte. Vi dà noia il volontariato; vi dà noia l'azione di solidarietà; vi dà noia perché non è nelle vostre corde, perché volete la tensione sociale, perché volete una società conflittuale dove si combatte per sopravvivere.

all'oscuro dei parlamentari, nel bel mezzo della notte ci volete far approvare. Però, signor presidente Conte, io ho un dubbio che le voglio rivelare. Perché lei fa tutto questo?

Lei sta affondando questo Paese! Lei vuol negare il futuro a questo Paese! Lei sta facendo una manovra pericolosa, che pregiudica lo sviluppo di questo Paese, che accentuerà la crisi e le difficoltà di questo Paese, avendolo fatto inginocchiare come non mai di fronte alla Commissione europea! Chiedo scusa, Presidente, ma dopo tante situazioni complicate in questi giorni, le chiedo ancora due minuti, che ha concesso a tutti. Signor Presidente

i suoi uomini, mi permetta, i suoi manipoli che sono venuti in Parlamento a umiliare il Parlamento su suo mandato. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il ministro Fraccaro è venuto a determinare il blocco della discussione nelle Commissioni e non viene un Ministro a caso. Viene perché il Presidente del Consiglio lo manda per impedire la discussione all'interno delle Aule parlamentari. Credo che la vergogna debba ricoprire il vostro il vostro volto in una serata triste per il nostro Paese e per la nostra storia. Concludo, signor Presidente: i tempi di questa discussione parlamentare sono stati questi per vostra volontà. E concludo, anche per rilassarci un pochino, con le parole di un autore che a noi abitanti dell'Appennino sono molto care e molto caro è questo autore: «Voi tenetevi le ghiande, lasciateci le ali». Le ali per volare di nuovo con questo Paese, che noi del Partito Democratico amiamo, nel quale crediamo e per il quale continueremo a combattere difendendolo dalla vostra politica scellerata.

onorevoli senatori, onorevoli senatrici, membri del Governo, intanto un ringraziamento va a tutti i membri della Commissione bilancio, a partire dal Presidente, che sono qui da più di dieci giorni a discutere. a portare avanti gli emendamenti, molti dei quali sono contenuti nel maxiemendamento, a testimonianza che il Parlamento ha discusso della manovra economica.

Eravate quasi certi della procedura di infrazione e l'abbiamo scongiurata. Queste previsioni nefaste ci fanno pensare, se è vero che la regola è «non c'è due senza tre», che la nostra economia crescerà nel prossimo anno. M5S)*. Compito della maggioranza è mettere in evidenza le note positive della manovra economica. Partiamo dalla famiglia,

modo, aumentiamo gli incentivi per gli asili nido, confermiamo il *bonus* bebè, rendiamo strutturali quelle misure fondamentali per aiutare le famiglie, per una ragione molto semplice: è dalle culle che dipende il futuro del nostro Paese. Sono previsti, come è stato detto, fondi anche per i disabili e i non autosufficienti. Nelle scorse manovre si doveva sempre rincorrere io ero in Regione Lombardia, ma chi era in Regione anche in altre parti d'Italia lo sa benissimo - i tagli: dal trasporto ai disabili al Fondo per la non autosufficienza. No, questa volta abbiamo 100 milioni di euro in più sul Fondo per la non autosufficienza; 100 milioni in più sul fondo per i disabili; 100 milioni per il trasporto dei disabili, perché per noi noi gli ultimi non sono solo gli immigrati. Parliamo delle imprese. Ci è stato detto che abbiamo aumentato le tasse perché sono andati a vedere una tabellina sulla manovra e dicono di aver visto 5 miliardi di euro in più nel 2019.

la riconferma di buona parte del pacchetto Industria 4.0, a testimonianza che quando si governa seriamente non si buttano via le misure che hanno fatto i Governi precedenti. Il raddoppio della detraibilità dell'IMU sui capannoni (dal 20 al 40 per cento) va proprio nella direzione dei tanti industriali imprenditori che hanno sofferto quella tassa che è stata messa non certo dal nostro Governo.

cento; poi portata nel 2020 fino a 100.000 con la tassazione al 20 per cento) è poca cosa: partite IVA, professionisti, artigiani, commercianti; tra l'altro c'è anche la cedolare secca per gli affitti proprio per aiutare gli esercizi commerciali in difficoltà. Ebbene, la misura è stata snobbata, non considerata, sminuita,

noi li aiutiamo. Certo che si può fare di più, ma è il primo anno; non è che si può fare tutta la *flat tax*. Lo avete detto voi che non si poteva fare in un anno solo, e adesso vi lamentate perché abbiamo dato solo l'avvio? Mettetevi un po' d'accordo anche tra di voi. piccoli professionisti che non hanno mai vissuto con i sussidi dello Stato, sia ben chiaro.

sia questo il vero partito del PIL - quei piccoli e medi imprenditori che, grazie alle misure che abbiamo inserito nella manovra, cominceranno ad aprire i cantieri per mettere in sicurezza nei nostri territori scuole, ospedali, tribunali, ponti, strade; L-SP-PSd'Az e M5S)*. Del resto, come facciamo a prendere lezioni sugli investimenti da chi ne ha messi 4,5 miliardi l'anno scorso e alla fine ha speso zero? Noi invece aiutiamo i Comuni: un miliardo vale solo l'aver sbloccato l'avanzo di amministrazione, 250 milioni alle Province tanto bistrattate (poi ci lamentiamo che ci sono le scuole che vanno a pezzi); non va dimenticato il *bonus* per gli enti locali (400 milioni inseriti nel maxiemendamento, che costituiscono un sostegno e un aiuto ai Comuni fino a 20.000 abitanti); lo sblocco dei finanziamenti che ci ha ricordato bene il sottosegretario Garavaglia

non solo non ci sono i tagli, ma addirittura gli diamo una mano, aiutiamo il nostro territorio. Ha ragione chi ha detto in quest'Aula - sempre, se non ricordo male, il sottosegretario Garavaglia - che mentre in Francia ci sono i *gilet* gialli, qui da noi ci saranno i *gilet* arancioni per tutti i cantieri che verranno aperti presto e questo farà prodotto interno lordo, questo muove l'economia. E poi arriviamo, *dulcis in fundo*, ovviamente alla quota 100, tanto vituperata dai membri della minoranza: con questa misura possiamo dire che si è davvero concretizzata

poco dopo le elezioni, la Commissione europea è intervenuta per dire che non si poteva toccare la riforma Fornero, perché la nostra spesa pensionistica era troppo alta. Questo era il monito, l'intimazione della Commissione europea.

che ha dovuto ammettere che l'Unione europea non mette in discussione la riforma delle pensioni che spetta al Governo italiano M5S)*, riconoscendo quella sovranità nazionale tanto indigesta a chi parlava di crisi indotte per costringere gli Stati a cedere la sovranità nazionale. Noi ce lo ricordiamo. *(Applausi dai

che oggi se c'è qualcuno che deve battere la ritirata, e noi consigliamo che sia silenziosa perché siamo buoni, sono coloro che hanno approvato la sciagurata riforma Fornero. Voi dovete battere in ritirata. E tutti quei partiti che l'hanno votata, altro che sconcerie su questa manovra. Ricordiamoci in passato cosa è successo e prendiamoci tutte le responsabilità.

e faremo di tutto sempre per il bene del Paese.

Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, credo che la giornata di oggi rappresenti e abbia chiuso purtroppo un percorso, una procedura che ha mortificato il Parlamento, nella sua massima espressione di rappresentanza del popolo italiano, sia in quest'Aula sia nel percorso della Commissione. Quindi, ha mortificato proprio quei cittadini che frequentemente vengono citati. Colleghi, io sono membro della Commissione bilancio e, unitamente ad altri colleghi, ho vissuto questi quindici in un dibattito anche aperto sui tanti temi di questa norma frastagliata formata da centinaia di commi, ma anche misurando nell'opposizione e nella maggioranza - anche se ufficialmente non si dichiara - uno stato di frustrazione rispetto al ruolo che il Parlamento della Repubblica, come massima espressione, deve avere.

tante questioni, alcune promesse, tanti tradimenti. Un provvedimento frastagliato, pieno di contraddizioni, senza un disegno politico, come ha avuto modo di dire nei vari interventi della giornata di ieri il presidente del nostro Gruppo Bernini, senza un disegno del Paese. Più soldi da una parte, più soldi dall'altra, più soldi presi a chi lavora duramente o a chi ha lavorato e gode di pochi euro di pensione. L'orgoglio dei poveri,

di molte famiglie che vivono con la cosiddetta pensione minima, di molte famiglie che non riescono a pagare tasse e tariffe della loro casa. Noi crediamo in un Governo che debba dare l'esempio e l'indirizzo, ed è giusto che chi ha la maggioranza governi e lo faccia.

Credetemi, non è per fare demagogia: la speranza dei giovani è anche la speranza delle loro famiglie, quindi anche di tutti quegli anziani che, nella società attuale,

L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea. I motivi dei ritardi sono stati imputati alla trattativa e al tira e molla con l'Unione europea. L'Italia - dicevo - è un Paese fondatore; chi vi parla e il Gruppo da cui parlo un Gruppo che dice e che ha detto più volte in quest'Aula che è giusto discutere con l'Unione europea, è giusto trattare, ma, da Paese fondatore, è giusto anche discutere le regole. Quindi si abbia il coraggio, come Paese, di rendersi conto che le regole di vent'anni fa non sono più applicabili oggigiorno, salvo la convenienza di altri Paesi e di altre Nazioni. Uso il termine «Nazione», e lo uso anche orgogliosamente. Il Governo non Il Governo non può usare l'Europa per danneggiare i propri cittadini, perché si ferma alla parte di trattativa nell'ultimo momento; è questo che noi imputiamo al Governo.

con una forma che non si sa ancora identificare: i 780 euro, con un modello che non conosciamo. Nel contempo si mortifica l'altra gente, quella che lavora. Forse Forse quelli è necessario invece prenderli per mano, accompagnarli e portarli a lavorare, non a ricevere il contributo elettorale. Quale democrazia abbiamo, se obiettivo del Governo non è più il bene del popolo, bensì l'esercizio alla punizione di chi non sta nei vostri sogni o nei vostri interessi, ma solo nella vostra convenienza elettorale? Questa è la questione Noi vorremmo e saremmo orgogliosi di opporci a una manovra di Governo che, diversa dal nostro pensiero e diversa da come la vorremmo fare noi, fosse almeno una manovra con un disegno di Paese, non un contratto. I temi, i grandi temi sono certo il reddito di cittadinanza, già trattato e che, come dicono molti di noi, è un insulto, un modello di propaganda del momento, certamente rispetto

abbiamo contrapposto l'ipotesi che non era possibile. Oggi la rivede all'1 per cento, ben 9 miliardi in meno; 9 miliardi sono 300.000 posti di lavoro, 300.000 famiglie. Siamo un Paese che ha bisogno di infrastrutture e di mantenere quello che ha. Noi apprezziamo positivamente quanto il sottosegretario Garavaglia ha espresso in quest'Aula e quanto

Ma non possiamo che rimarcare il passo indietro sugli investimenti e - permettetemi, io vengo dal Nord - il fatto che si fermino investimenti già avviati, quali la TAV. Il Governo ora annuncia che farà un miliardo in più di dismissioni. Una precisazione: se sono una finzione, si rischia di usare male il risparmio postale degli italiani.

2012 e gli effetti sono stati probabilmente pari a quasi 100 miliardi di minori introiti per lo Stato. Voi direte:

del 2019. Noi avremmo voluto anche prendere in considerazione un intervento sull'IVA, ma con contestuale valutazione della riduzione, anche se non proprio sotto dell'IRPEF. Questo era il disegno del centrodestra e questo è il disegno che speriamo i colleghi della nostra coalizione elettorale (e attualmente della vostra coalizione di Governo) portino avanti. È una manovra d'azzardo, non solo per le tasse sui giochi,

che il Governo ha fatto su alcuni settori, come la sicurezza, non possiamo non rimarcare come non è apprezzabile la parte di politica economica che riguarda la politica sociale di questo Paese.

Signor Presidente, qualcuno voleva imporci una manovra con un rapporto *deficit-* PIL pari all'1,6 per cento, ma non ci è riuscito perché questa è una manovra scritta in Italia, *made in Italy*, e non è *made in Europe*

semplicemente perché conosce soltanto la grammatica dell'austerità e cari professori, cari oppositori, voi ormai parlate la stessa lingua dell'austerità, la stessa lingua dell'Europa, per questo non riuscite a capire questa manovra. la metà della sensibilità sociale che caratterizza questa manovra, oggi non vivrebbe la crisi sociale e popolare che è sotto gli occhi di tutti PD).* La rivolta dei *gilet* gialli è la rivolta dei nuovi miserabili, quelli schiacciati dall'austerità, i nuovi miserabili creati dal cortocircuito tra una globalizzazione senza regole, per la quale facevate il tifo, e il fanatismo mercatista e finanziario. Onorevoli colleghi, siamo andati a Bruxelles, sì, ma siamo andati per indicare una nuova rotta, che è la rotta sociale *(Applausi Chi ha creato la rottura sociale ora sta chiedendo scusa: Macron, il vostro nuovo *guru,* si sta piegando al volere del popolo, perché quando il popolo impone una trattativa ha già cominciato a vincere. Reddito di cittadinanza e quota 100 sono l'opposto di quello che l'Europa avrebbe voluto. Altro che dettatura; avere una stabilità finanziaria, senza avere una stabilità sociale, significa guidare ad alta velocità, a fari spenti nella notte, vuol dire andarsi a schiantare e questo noi per l'Italia e gli italiani non lo vogliamo. Cara opposizione, cari oppositori, un giorno ci ringrazierete per avere protetto l'Italia dalle tensioni sociali, perché un Paese in subbuglio incrina qualsiasi equilibrio finanziario. Questa manovra, se la dovessi e la potessi raffigurare con un'icona, la raffigurerei come una mano tesa, che tendiamo a chi cerca di rialzarsi, a chi cerca un conforto. Che cosa è il reddito di cittadinanza, che tanto non piace a questi signori, se non un'altra *chance* che offriamo? Potete giocare con le sottrazioni magiche, ma l'unico numero è 7,1 miliardi per il reddito e le pensioni di cittadinanza. Voi ci avete lasciato 5 milioni di poveri; non ce lo possiamo dimenticare, non è tana libera tutti.

Ci avete lasciato una platea di pensionati invisibili che vanno a raccattare la merce in fondo alle periferie dei mercati e questo è profondamente ingiusto, cari signori. Ci avete lasciato questa platea di pensionati invisibili e noi gli daremo la pensione

una riforma delle pensioni, la famigerata riforma Fornero, ingiusta, crudele e iniqua. Noi la cambiamo, anche se all'Europa non piace. Voi avevate scritto sotto dettatura dell'Europa quella riforma, noi la cancelliamo con il volere del popolo. Non avete mai toccato le pensioni d'oro, forse per non urtare la sensibilità dei vostri amici, e ci tocca sentire in televisione il piagnisteo di gente che dice che non sa più come vivere

Ci avete consegnato una sanità sempre più lontana dai cittadini e con gli investimenti previsti in questa manovra noi ridurremo drasticamente i tempi di attesa e faremo altre cose per puntellare una sanità che deve essere pubblica. E che dire dei risparmiatori truffati. Ci voleva questo Governo per mettere un miliardo e mezzo in un fondo per risarcire i truffati dalle banche; volte di più di quello stanziato precedentemente. Avete il coraggio di negarlo? Voi inciuciavate con i banchieri, noi risarciamo i risparmiatori. E diamo ai risparmiatori la possibilità di rivalersi anche verso la Banca d'Italia, la Consob e le banche, perché noi non abbiamo amichetti da difendere, da coprire o parenti da tutelare. Così come del resto non abbiamo avuto fuori dalla porta i lobbisti che chiedevano di cambiare la manovra. Dicevate che non c'erano investimenti; abbiamo previsto un fondo importante per realizzare opere che interessano la quotidianità dei cittadini. Cari cittadini, pretendete dai vostri sindaci le opere che davvero chiedete, dalle strade alla messa in sicurezza degli edifici scolastici o altre infrastrutture.

e non per gli appetiti di amichetti o di cartelli di imprenditori, anche perché con lo spazza corrotti la mangiatoia è chiusa.

PD).* Abbiamo fatto la *flat tax* e abbiamo cominciato il percorso di revisione fiscale. Lo abbiamo fatto per una platea di piccolissimi imprenditori e per le partite IVA.

Questa è una manovra tutta scritta in Italia; porta il marchio del *made in Italy*. Questa è la manovra del cambiamento e per questo il Gruppo MoVimento 5 Stelle dice sì. Per favore, tirate giù i cartelli.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione

Bongiorno, Bossi Umberto,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

Onorevoli colleghi, poiché sono stati esaminati tutti gli articoli al disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile. La 5a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea. In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta. *(La seduta, sospesa assegnazione** Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato la "Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della prima sezione.

si tratta della Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato al disegno di legge di Si segnala che la suddetta Nota aggiorna i valori contabili dell'articolo 16 (Totale generale della spesa) del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche: ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2019-2021 in termini di competenza e di cassa; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1 ) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a 14). Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli. I prospetti sono organizzati per unità di voto e gli allegati tecnici presentano l'intero bilancio dello Stato e con evidenza delle unità e dei capitoli che hanno subito variazioni per effetto degli emendamenti al disegno di legge; le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la Sezione I e la Sezione II. una nuova finestra"). Passiamo dunque alla votazione della Seconda Nota di variazioni. Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle. Indìco la votazione